grazie a tutta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

recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali"

Faccio rilevare che questo tipo di attività non può sconfinare entro certi limiti di carattere anatomotopografico relativi proprio al distretto di interesse della disciplina di odontoiatria. del 1985, che si va a modificare, prevede che formino oggetto della professione di odontoiatria le attività inerenti alla diagnosi e alla terapia delle malattie e anomalie congenite ed acquisite dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti. Sebbene questo possa rappresentare un problema di carattere molto tecnico, vorrei evidenziare a tutti i membri del Parlamento che nel momento in cui si dà all'odontoiatra la possibilità di agire non solo sul terzo inferiore e sul terzo medio della faccia (cosa alla quale sono favorevole), ma anche sul terzo superiore, si sta commettendo una irregolarità grossolana. il terzo superiore della faccia, che comprende le orbite e la fronte, non è all'interno dello splancnocranio, che è la parte della faccia

nel terzo medio della faccia. Se si fa uno sconfinamento nel terzo superiore della faccia - e prego i colleghi di ascoltarmi attentamente

si prende la responsabilità di un provvedimento che è completamente contrario a ciò che è scritto nei testi di anatomia topografica. Ripeto che si tratta semplicemente di una correzione che deve essere apportata necessariamente: non c'è possibilità di prendere in esame un distretto della faccia

firma per contribuire a questa piccola modifica, che consentirà di avere un provvedimento veramente efficace ed utile.

dopo una lunga maturazione alla Camera dei deputati. Devo dire che innanzi tutto la modalità con cui sono stati organizzati i lavori ci porta assolutamente ad un giudizio negativo. Il Senato non è riuscito di fatto ad esprimere nelle Commissioni pertinenti un parere articolato né ad intervenire sugli emendamenti fortemente modificativi del testo che sono maturati alla Camera dei deputati. Comincerei dicendo questo, visto che parliamo

carovita, l'inflazione, le bolle speculative sui prodotti di prima necessità, le questioni dirimenti riguardanti il lavoro e i salari lo hanno reso infatti un anno non facile per le famiglie italiane. In questo Parlamento possiamo dire che ormai la luna di miele del Governo è finita, il momento delle riforme non c'è stato e non è arrivato. Non è arrivato con questo decreto-legge in cui noi avremmo immaginato la possibilità di intervenire almeno chirurgicamente, mettendo in campo alcune riforme di sistema che pure erano state annunciate *in primis* in materia di sanità, su cui poi farò

che la copertura del *recovery fund* è sulla nostra testa un elemento di garanzia che permette al nostro prodotto interno lordo di reggere le bordate della contemporaneità che arrivano dal lato della riorganizzazione dei sistemi bancari e delle questioni legate ai tassi di interesse.

il richiamo all'Italia non solo sulle questioni storiche su cui veniamo sempre richiamati (il *deficit*, la produttività del nostro sistema lavoro e la mancata applicazione delle riforme), ma anche sulla mancata attuazione o implementazione delle riforme che sono previste e che sono proprie del PNRR. Tra di esse, vi sono le questioni su cui la maggioranza si è particolarmente concentrata in questi mesi, e cioè il tema delle concessioni demaniali, che è stato l'oggetto principale del dibattito politico concreto nel nostro Paese, e i temi legati alla concorrenza, che sono ancora tutti là e non si sa se e quando arriveranno. Dall'altra parte, vi è poi un richiamo non banale al tema del fisco, che non è che non si incroci con questo decreto-legge; si incrocia eccome, si incrocia eccome, per com'è impostato il decreto, con una serie di operazioni *spot*, ma soprattutto rispetto a quello che è previsto o che pare prevedibile nei prossimi anni dal richiamo che ci è stato fatto sull'estensione della *flat tax*, che viene definito iniquo e crea confusione, all'altro pezzo di riforme su cui siamo stati richiamati, cioè la paventata riforma dell'autonomia differenziata, che pure mette a rischio il sistema del bilancio pubblico oltre al tema della funzionalità del nostro ordinamento. Siamo quindi in un momento in cui le misure messe in campo o sul piatto dal Governo destano qualche perplessità non soltanto nelle opposizioni, ma direi anche negli osservatori europei, non tanto per un ragionamento politico, quanto sul tema della nostra stabilità finanziaria e della nostra capacità di ripagare il nostro debito quando ci verrà richiesto,

100 o 200 miliardi, sono state soltanto l'ennesima bandierina politica presentata agli italiani. Poi non ci meravigliamo che gli italiani si astengano, non vadano a votare e vengano presi da una sorta di sconforto per cui pensano che nulla possa cambiare. Il primo nostro dovere ce l'abbiamo qui, almeno con un richiamo alla realtà.

ristoro dall'aumento del gas, ma vengono rimessi gli oneri in bolletta che erano stati cancellati. Questo vorrà dire che a breve, quando questa misura, che è temporanea, ci ritroveremo che da una parte ci danno e dall'altro ci tolgono. Speriamo solo che nel frattempo saremo riusciti a mettere in campo le misure per la transizione ecologica e che quindi avremo altre misure di approvvigionamento per quanto riguarda l'energia, che ci permettano di tenere contenuti i

Purtroppo sulla sanità in questo Paese stiamo facendo un esercizio poco utile, nel senso per tre anni si è parlato tutti i giorni non di sanità, ma di epidemia,

e sulle spese sanitarie e il grandissimo tema legato al personale sanitario. Il Ministro aveva promesso che in questo decreto-legge si sarebbero affrontate questioni che erano state rinviate anche dalla legge di bilancio e che quindi non erano state affrontate: *in primis,* il tema del pronto soccorso e dell'urgenza, la remunerazione e la stabilizzazione del personale, e i temi legati alla formazione specialistica e al cosiddetto

messa una fine alla questione dei gettonisti, per poi tornare indietro; abbiamo avuto l'annuncio che avremmo risolto il tema dell'aumento degli stipendi e delle indennità per gli operatori del pronto soccorso per tutto l'anno, e siamo tornati indietro. Ma le riforme dove sono? Il Governo quando ce le presenta, queste riforme? Quando avremo una riforma del personale sanitario? Quando avremo una riforma dell'arruolamento e della formazione degli infermieri? Anche sulla parte legata all'articolo 15, quanto alla necessità di assumere personale straniero, ad esempio, perché abbiamo una carenza in alcune aree del comparto, non c'è nulla di strutturato. Non c'è una proposta di riforma che ci permetta di riorganizzare il sistema rispetto alle emergenze che ci sono ora sul territorio. Penso all'Emilia-Romagna e al rischio biologico relativo alla depurazione delle acque, all'antitetanica e a quello che sta accadendo nell'emergenza

i termini degli elenchi, lo facciano pure, ma rispettando i criteri che vanno contro l'abuso della professione sanitaria e che quindi sono a tutela della sicurezza dei pazienti

fosse, mettendo seriamente a rischio l'organizzazione complessa di questo settore. Tutti gli altri operatori del comparto, che rientrano nelle professioni sanitarie, è come se non esistessero ed è stato fatto un provvedimento, che in questo caso non

non fa bene a nessuno, non fa bene alle istituzioni che rappresentiamo, non fa bene allo Stato in generale e neanche alla maggioranza, perché poi i problemi sul campo sono tantissimi e molto complicati.

la conversione del provvedimento in esame, che ci vede senz'altro favorevoli, perché tiene conto di una rilevante consistenza di esigenze del Paese, in economia e in sanità, anche sul versante dell'emergenza e urgenza, recependo una serie di necessità che ci hanno visti da tempo impegnati sull'argomento, ci lascia però un amaro in bocca e un profondo rammarico, perché non si è voluto - o potuto - inserire un piccolissimo emendamento,

la soluzione messa a punto con il coinvolgimento proattivo delle casse previdenziali, di modestissimo impatto economico del tutto irrilevante nel bilancio dello Stato, per arrivare a riconoscere finalmente un giusto, seppur tardivo, ristoro ai medici vittime del Covid, prioritarizzando la categoria più colpita, ovvero i medici, rimasti senza alcun indennizzo in forma assicurativa, che durante la prima fase della pandemia hanno patito menomazioni permanenti e i familiari di quei medici deceduti, in alcun modo ristorati. Sono convinta della bontà della proposta, che continueremo a prospettare con tenacia e pervicace determinazione, perché non sono solo le celebrazioni del 18 marzo di ogni anno che ci devono far ricordare le vittime del Covid, ma una società più giusta, quale quella a cui dobbiamo tendere, deve saper onorare, con la concretezza e la riconoscenza, chi ha avuto il coraggio di agire il coraggio di agire per salvare altre vite. Ed è per questo che sono convinta che col tempo tutti ce ne convinceremo, a meno che non ci sia una pregiudiziale, perché è chiamato emendamento Cantù; che si chiami come meglio pare, purché ci sia semaforo verde. Io non cerco visibilità. modo, in questi ultimi tre anni, abbiamo elaborato un riordino della medicina territoriale per il rilancio del ruolo del medico di famiglia, valorizzandolo e responsabilizzandolo, anche in memoria di chi spontaneamente ha dedicato se stesso, fino al gesto estremo, per salvare altre vite. Ed è anche per questo che la professione del medico di medicina generale, che è stata la più colpita in emergenza pandemica, pandemica, dal nostro punto di vista non solo merita di essere giustamente ristorata, ma dovrà essere proattivamente rilanciata e riqualificata in chiave ordinamentale, così come abbiamo previsto nella risoluzione di accompagnamento al Documento di economia e finanza, perché ci si è resi conto di quanto il medico di famiglia sia una figura determinante nel nostro sistema sanitario.

aggiornamento normativo che darà certezza di continuità e di prossimità di cura a tutti quei bisogni che non richiedono ospedalizzazione, in chiave universalistica ed equiaccessibile.

in effetti, l'aiuto sulle bollette è riferito a soli quattro articoli su 24. Di questo decreto noi non salviamo quasi nulla, ma tornerò sul punto. Vorrei sottolineare un aspetto: deputati, in un primo momento, avevate inserito la stabilizzazione dei ricercatori precari nella sanità pubblica, una categoria tenuta per decenni in una condizione di precarizzazione sistematica, per poi stralciare, dopo averli approvati in Commissione, gli emendamenti per assenza di copertura. Quindi, anche la maggioranza probabilmente non lo ha chiaro, perché non si può dire che non si è voluto Non si è potuto discutere, né in 10a Commissione, né tantomeno nelle Commissioni riunite. Sostanzialmente è un provvedimento chiuso, che è arrivato in questo modo: prendere o lasciare. Avete scelto di confermare l'indennità dei medici e degli infermieri dei servizi di emergenza e urgenza e di estendere il ricorso ai gettonisti non soltanto ai servizi di emergenza e di urgenza ospedaliera, come si indicava nel testo iniziale del decreto, ma anche ad altri reparti. L'articolo 10 permette alle aziende del Servizio sanitario nazionale di procedere all'esternalizzazione dell'affidamento a terzi di servizi medici, anche prorogando i contratti in corso di esecuzione per tutte le specializzazioni. la stretta non si applicherà ai contratti derivati da procedure di affidamento che prevedono il conferimento di attività ai servizi sanitari in gestione agli operatori economici per la riqualificazione delle strutture sanitarie e dei presidi ospedalieri. Il fatto è che sappiamo benissimo qual è la situazione di partenza: medici e infermieri in affitto senza essere nemmeno iscritti all'albo professionale;

Allo stesso tempo, i dati ci dicono che mancano 300.000 medici, soprattutto ospedalieri, ma c'è un dato che dovrebbe preoccupare tutti noi: ogni giorno sette medici vanno via dal sistema pubblico, si dimettono. Il fenomeno è aumentato del 39 per cento nell'ultimo anno.

del fatto che aspettano mesi e anni per un esame diagnostico? Che non ci sono i soldi? O che li abbiamo spesi per pagare i gettonisti? Di fronte a tutto ciò, la maggioranza mette nero su bianco un'ulteriore spinta alla privatizzazione. Da un lato, l'autonomia differenziata che, va verso un regionalismo asimmetrico, quindi di fatto vi è la negazione del senso stesso del *welfare*; dall'altro, vi è un tetto di spesa che blocca le risorse per assumere personale e per rinnovare i contratti collettivi nazionali di lavoro. Oggi, di fatto, in Italia chi può, perché

che ci sono 4 milioni di persone in questo Paese che rinunciano alle cure per motivi economici. Insomma, il diritto alla salute pubblica e gratuita per tutti sta scomparendo. Credo che questa sia l'emergenza nelle emergenze e che tutti noi dovremmo farcene carico. Ecco spiegato perché rinunciare a intervenire sui gettonisti è solo rinunciare a intervenire sui gettonisti è solo l'altra faccia di questa medaglia: la carenza endemica di medici richiederebbe interventi strutturali, volti a ripensare l'assistenza mettendo al centro la la persona, la comunità e il territorio; richiederebbe la valorizzazione di tutte le figure professionali che si spendono per il Sistema sanitario nazionale; richiederebbe il coraggio di superare i limiti che non permettono di assumere in modo strutturale il personale; richiederebbe di stanziare almeno il 7 per cento del PIL nazionale

Avete deciso di varare uno scudo penale, l'ennesimo condono per gli evasori, inserito all'ultimo secondo. La maggioranza infatti depenalizza l'omesso versamento, perché i 12 condoni della legge di bilancio evidentemente non sono bastati. bastati. In sostanza, si va in questa direzione. Sarebbe ora che questo Governo prendesse in mano le questioni vere del nostro Paese: la tenuta della sanità pubblica, l'attuazione dei progetti finanziati con il PNRR, la valorizzazione del personale sanitario, senza dimenticare i ricercatori precari e la lotta all'evasione fiscale, smettendo di strizzare l'occhio agli evasori. Insomma, si premiano gli elusori e gli evasori, nemici del *welfare*, e si è sordi nei confronti della stragrande maggioranza delle persone. Infine, voglio sottolineare l'unica cosa che ritengo positiva di questo decreto-legge: all'articolo 24, comma 2, la costituzione di un fondo

prima di tutto bisogna dire che il decreto-legge in esame prosegue con la politica di aiuti ai più deboli già messa in campo da questo Governo. alle misure contenute nel decreto, oltre alle tematiche energetiche, affrontiamo i rincari delle bollette di energia e del gas, la tematica della sanità e quella degli adempimenti fiscali. Le tante articolate misure contenute del decreto sono sostenute da risorse economiche per 5,5 miliardi di euro per tutto il 2023. economie di bilancio che dimostrano la gestione molto prudente delle finanze che ha consentito, a pochi mesi dalla legge di bilancio del dicembre 2022, di trovare nuove coperture finanziarie alle misure che il Governo riteneva fondamentali per sostenere il Paese. Pesano Pesano ancora, infatti, gli effetti della crisi energetica internazionale, che si fanno sentire soprattutto su alcuni nuclei familiari più fragili. Il Governo prosegue, quindi, in questa politica di sostegno, perché è convinto, con la sua maggioranza, che solo sostenendo le famiglie italiane può tenere insieme tutto il tessuto sociale e la propria economia. L'economia italiana cresce con valori superiori a quelli degli altri Paesi europei e questo conferma che le politiche economiche adottate sinora sono state quelle più appropriate. Anche a dicembre, gran parte delle risorse è andata a sostenere famiglie e imprese, evitando i danni del caro energia. Ora - come detto - si prosegue nella stessa direzione, modellando molte misure di sostegno al nuovo quadro economico. Allo stesso modo, nel decreto-legge si affronta il tema importantissimo della spesa farmaceutica e di come procedere con regole che siano chiare per i fornitori, per le Regioni e per lo Stato. Si affronta, però, anche il tema del funzionamento dei pronto soccorso, il problema fondamentale della presenza di questi presidi sui territori, che purtroppo non riescono più a garantire quello straordinario e fondamentale servizio ai cittadini. È un tema che conosco bene e che ho già affrontato, presentando interrogazioni e durante il *question time*, per tutelare i presidi sanitari della mia terra, la Campania, è il problema relativo alla presenza dei medici e del personale sanitario, che viene risolto introducendo norme di buon senso. Le persone in prima fila nella sanità devono essere retribuite in modo adeguato per il loro lavoro, per la loro abnegazione e per la loro disponibilità a lunghi straordinari. In tal modo, dovrebbe essere superato anche il problema dei cosiddetti gettonisti. Allo stesso tempo deve essere garantita, a chi lavora nell'interesse degli altri, la propria incolumità. Non è più tollerabile che chi lavora e interviene per curare un malato rischi di venire aggredito e malmenato dai parenti. Ora si potranno istituire dei posti di polizia a presidio delle strutture ospedaliere, per proteggere medici e infermieri in prima linea. Da ultimo, vorrei sottolineare l'importanza della messa a punto delle regole relative agli adempimenti fiscali. Come abbiamo già detto, è ancora un momento critico per la nostra economia, seppure essa abbia reagito meglio degli gli altri Paesi europei. Dietro la creazione di prodotti e di ricchezza ci sono spesso piccoli imprenditori, partite Iva che devono affrontare il tema degli adempimenti fiscali. consentire, dunque, loro di dilazionare i pagamenti, di non essere messi alla gogna per aver saltato un pagamento; di fare in modo che, grazie a uno Stato meno patrigno, possano adempiere alle loro scadenze e ripartire. Questa ci pare un'altra ottima previsione di questo decreto. Si potranno dilazionare i pagamenti sanitari, con uno Stato più amico verso chi vorrà contribuire con il proprio lavoro a far crescere la nostra economia. Insomma, questo Governo ancora una volta si fa carico delle problematiche degli italiani che lavorano e producono, mettendo in campo norme mirate e risorse adeguate per sostenerli. Il decreto segna, quindi, ancora un passo in avanti nell'azione di Governo, che noi sosteniamo in modo convinto.

Per questo voteremo contro questo provvedimento, perché va proprio nella direzione sbagliata, quella che non dovremmo prendere. Stiamo solo perdendo tempo e stiamo complicando

investe nella digitalizzazione e nell'ammodernamento della propria attività o propria impresa. Siamo d'accordo su una riduzione delle tasse, ma con un fisco premiante

state incentivando fonti fossili che andate a cercare nel globo terracqueo, in tutti i Paesi, come l'Algeria. Cercate fonti fossili da incentivare ed è sbagliato, perché quelle sono fonti che arrivano dall'estero: possono aumentare i prezzi, possono chiudere i rubinetti. Voi dovete invece parlare - come

è più comprensibile, perché non ho questo tipo di narrazione, ma posso imparare, con la speranza che anche voi della maggioranza mi ascoltiate. Noi potremmo parlare di patriottismo energetico: imprese e famiglie che si immolano per dare sovranità energetica alla nostra Patria.

Capite che quella è l'energia interna, l'energia *made in Italy*, l'energia tricolore? È l'energia che ci può assicurare sia stabilità nei prezzi, sia fornitura per i prossimi anni, ma che

avremmo avuto nei prossimi anni 40 miliardi di energia *made in Italy*. Questi sono gli investimenti che dobbiamo fare e non perché ce lo chiede l'ambiente, ma perché sono convenienti dal punto di vista economico.

sicurezza energetica, ambiente. Cerchiamo almeno di fare un piano strutturale per le fonti alternative partendo da leggi che già esistono. In Puglia, ad esempio, il reddito energetico in questi giorni sta consentendo a decine, centinaia di famiglie di avere un impianto fotovoltaico gratuito. Come? Con un meccanismo semplice, come vi ho detto. Se noi investiamo 10 miliardi sul fotovoltaico da installare su tetti delle imprese e delle case delle famiglie, ne produrremo 40-50, in base al territorio.

capire che il mondo è cambiato, i problemi sono cambiati, come lo sono le tecnologie. Avete una politica vecchia, ormai superata, che purtroppo farà sì che in questi cinque anni

In questi cinque anni si decide il futuro dei prossimi trenta. E, se non lo capite e continuate con questa politica vecchia, che non fa altro che aumentare i danni e ritardare la

per chi investe in efficienza energetica, in sicurezza del Paese, in digitalizzazione e rinnovabili. Questo è il fisico che vogliamo: meno tasse per chi investe nel futuro.

al *payback* sui dispositivi medici, che a mio avviso va definitivamente superato. E cerco di argomentare perché bisogna trovare una soluzione definitiva che superi questo strumento che ha dimostrato di non funzionare. fu introdotto anni fa dai Governi di sinistra pensando di fare cassa, ma non si è mai riusciti a farlo partire e adesso sta dimostrando di tirare la corda, di non funzionare. qualche esempio: innanzitutto è profondamente iniquo, tant'è che nel decreto-legge è stato previsto più di un miliardo per aiutare le Regioni che non sono riuscite ad applicare questo strumento. L'obiettivo del *payback* - per chi non lo sapesse - è porre un freno al consumo dei dispositivi medici, prevedendo un tetto: se sfori il tetto, pagano le Regioni e i produttori. Questo, però, implica una capacità di programmazione che non c'è fino in fondo. Da qui l'iniquità. Abbiamo postato più di un miliardo: bene, si penserà che così abbiamo aiutato tutte le Regioni, ma non è proprio così. Sapete quanto va alla Regione Lombardia di questo un miliardo e 85 milioni?

è come migliorare la programmazione. Il Ministero della salute dovrebbe fare di più, dovrebbe aiutare maggiormente le Regioni a fare programmazione negli acquisti. Faccio due esempi:

Una ASL può fare una gara e comprare uno stent di ultima generazione, che addirittura, tramite sensori e un *software* collegato, consente di dare un avviso di un potenziale infarto

mettere un tetto economico, che non funziona per come è il mercato dei dispositivi medici, che è profondamente diverso da quello dei farmaci: più di 40.000 referenze, più di 40.000 prodotti, spesso con una componente di servizio difficilmente quantificabile.

La componente di servizio è difficilmente quantificabile, tant'è che in altri Paesi non si compra il prodotto in quanto tale, ma il prodotto più la componente di servizi;

all'aiuto al mercato, perché si facilitano davvero i produttori piuttosto che i distributori, i quali non fanno altro che commercializzare un prodotto, lucrando la differenza. poi prestare massima attenzione a non crearci da soli un tagliafuori rispetto agli altri Paesi che stanno correndo più di noi sulla tecnologia. Mi spiego: insistere sul meccanismo sciocco del *payback*

Spero di aver contribuito a portare un minimo di chiarezza su un argomento che è molto poco conosciuto dal Parlamento, ma che rischia di metterci

ho sentito affrontare - veramente solo accennare - temi molto importanti, come il *payback* e il costo dell'energia. Sono temi fondamentali, per cui non si può non iniziare questo intervento - come hanno già fatto alcuni colleghi prima di me, a cominciare dalla senatrice Lorenzin - lamentandosi e rammaricandosi per questo metodo. Io comprendo

aveva qualche elemento di angosciante preoccupazione e drammaticità in più di quella attuale. È difficile accettare che ci si possa trovare in condizioni in cui non si può mai discutere di niente, senza mai riuscire a confrontarsi su nulla. Ho ascoltato l'onorevole Garavaglia citare la Ferrari e la 500. Voglio dirgli mio avviso, con questo metodo non si costruisce né la Ferrari, né la 500. Voglio anche ricordare che l'onorevole Meloni definiva pannicelli caldi i 49,5 miliardi di euro che complessivamente il presidente Draghi mise sul decreto bollette; se quello era un pannicello caldo,

prendendo anche atto che ormai noi siamo a una forma di monocameralismo di fatto. Praticamente, quando un provvedimento viene discusso e affrontato in una Camera, nell'altra

della patologia, cioè di una pandemia violentissima. Sappiamo tutti e siamo consapevoli che la sanità sta attraversando una enorme difficoltà. Questo provvedimento è stato venduto e presentato come una sorta di grande riforma della sanità; in realtà dentro c'è al massimo - come detto da una mia collega alla Camera - qualcosa che assomiglia ad un *maquillage*.

preoccupano moltissimo. Nel DEF ci sono segnali di definanziamento; a partire dal 2025, il rapporto spesa sanitaria-PIL si attesterà

l'investimento nella spesa sanitaria e, rispetto alle previsioni di spesa sanitaria sino al 2026, il DEF 2023 certifica l'assenza di un cambio di rotta *post* pandemia. Potete continuare a dire quello che si sente ormai come una specie di litania che poi un giorno avrà - immagino - un punto di conclusione, perché arriverà un momento dal quale da lì in poi la responsabilità delle scelte

È stato detto in molti modi. In questo momento il Servizio sanitario nazionale corre davvero il rischio di superare il punto di non ritorno. I principi di universalità, di uguaglianza ed equità sono minati da criticità che compromettono il diritto costituzionale alla tutela della salute. Le liste di attesa costringono a ricorrere al privato, aumentano la spesa *out of pocket* e impoveriscono le famiglie, ma non possono essere spese sostenute da chi è già in una condizione di difficoltà.

Diteci come stanno le cose. Non vorremmo dover scoprire che anche le risorse destinate alla sanità stanno messe male. Le organizzazioni sindacali di categoria hanno detto che il decreto-legge in discussione contiene misure per lo più di ordine normativo e rigorosamente senza impegni economici. L'unico messaggio che - lo voglio precisare - consideriamo vagamente positivo è riservato ai soli pronto soccorso.

Il Ministro della salute è intervenuto più volte per dire che avrebbe anticipato l'indennità facendola partire dal gennaio 2023, ma questo in realtà non si è ancora verificato.

Non c'è alcuna considerazione per altre discipline che hanno problemi altrettanto gravi: anestesisti, chirurghi, professionisti della prevenzione primaria e coloro che prendono in carico i pazienti *post* acuzie.

un decreto-legge che in realtà non affronta davvero un problema che consideriamo e continuiamo a considerare drammatico. Su questo - e mi avvio a concludere - non posso non lanciare davvero un un appello a ripensare la questione della stabilizzazione dei ricercatori precari che lavorano negli istituti di ricerca e negli istituti zooprofilattici zooprofilattici sperimentali: sono giovani che vivono da anni con contratti a tempo determinato, senza alcuna possibilità di stabilizzazione. Vi voglio chiedere: voi che parlate di natalità e di famiglia come credete che un giovane possa pensare di pianificare una vita familiare quando in realtà si continua a dargli risposte che non prevedono per lui la possibilità di farlo? Sembra davvero il gioco della volpe e dell'uva. quindi a ripensare a queste misure e a rimediare. La nostra è davvero una bocciatura assoluta sia nel metodo che nei contenuti.

a nome del Governo, autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti né articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge n. 714, di conversione, con "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese

nuova finestra"). La Presidenza prende atto della posizione della questione di fiducia sull'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 34, nel testo identico a quello approvato dalla Camera dei deputati.

I rincari delle bollette di luce e gas infatti, sebbene in un contesto meno grave rispetto al passato, continuavano a mettere in grave difficoltà soprattutto l'anello più debole della catena del nostro tessuto sociale: le famiglie con i redditi più bassi e le nostre imprese, soprattutto quelle piccole e medie e le imprese artigiane. Oggi con questo provvedimento si dà una risposta concreta alle attese e ai bisogni di tanti italiani. La lotta al caro energia per questa maggioranza di centrodestra è sempre stata una

che ci apprestiamo oggi a convertire in legge. Ciò che ha fatto questo Governo in questo difficilissimo inverno va riconosciuto. C'è stata una strategia composta da più azioni integrate fra loro, non ultimo l'atteggiamento determinato e incisivo dell'Italia in sede europea, dove - come tutti noi sappiamo - si è giocata la partita per stabilire il prezzo massimo all'acquisto del gas. Il TTF (Title Transfer Facility) olandese è tornato a circa 30 euro per megawattora: un livello così non si vedeva da almeno due anni. Solo per renderci conto, il record venne raggiunto ad agosto con oltre 320 euro per megawattora. I numeri sono eloquenti: abbiamo invertito la rotta. Senza questa partita non avremmo mai fermato la speculazione che avrebbe continuato a sottrarre miliardi e miliardi dalle tasche dei nostri cittadini e delle nostre imprese. Questa strategia vincente è data anche da provvedimenti concreti, come quello oggi all'esame di quest'Assemblea. Usciamo dal 2022 con un'inflazione al 12 per cento e con l'incremento dei beni alimentari al 13 per cento. Quale criterio dovevamo utilizzare nel definire gli aiuti contro il caro energia? Non certamente quello di distribuire soldi a pioggia a tutti. Abbiamo fatto una scelta precisa e ponderata: concentrare la maggior parte degli sforzi sulle famiglie meno abbienti, perché questo succede in una famiglia; questo fanno un papà o una mamma: assicurare il proprio sostegno ai propri figli, ma dando la priorità a chi è più in difficoltà. Sostenere le fasce sociali più basse: non è questo che interessa teoricamente anche all'altra parte di quest'Aula, alla sinistra? Già, in teoria è così; i fatti ci dicono altro. L'opposizione vota no e pone censure rispetto a un provvedimento che ha alla base il principio dell'equità sociale, ovvero aiutare chi sta più indietro. Per le imprese, grazie a tutta la compagine governativa, si inaugura una nuova stagione, perché dietro un'impresa c'è lavoro. Ancora una volta le norme approvate pongono al centro il sistema produttivo per garantirne la competitività. L'economia reale, come ha detto il presidente Meloni pubblicamente, è il *core business* di questo Governo. Vogliamo uno Stato che sia alleato, e non avversario, delle nostre imprese. Questa è la visione condivisa che ci ha spinto con il cosiddetto decreto lavoro ad archiviare il reddito di cittadinanza, un sussidio che era pensato, purtroppo, per chi voleva stare a casa sul divano. Vogliamo creare lavoro, perché di questo hanno bisogno i nostri cittadini e le nostre imprese, da Nord a Sud. Tornando al provvedimento di oggi, sono diverse le misure previste, tutte molto importanti. Cito le più importanti: proroga e potenziamento del bonus sociale elettrico proroga del taglio IVA al 5 per cento per il gas metano per usi civili e industriali; azzeramento oneri di sistema per le utenze di gas; credito d'imposta per le impresa al 40, e al 45 per cento se nel primo trimestre 2023 hanno registrato un incremento delle bollette di luce e gas pari o superiore al 30 al primo trimestre del 2019; agevolazioni per le aziende agricole che fanno parte, non a caso, del settore primario, perché senza i nostri agricoltori che lavorano la terra non c'è futuro per nessuno di noi; incentivi fino a 200.000 euro per le *startup* che sviluppano progetti legati, ad esempio, alle rinnovabili. Mi preme evidenziare che, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera, sono stati approvati emendamenti emendamenti particolarmente rilevanti, che riguardano la vita concreta dei nostri cittadini. Mi riferisco, ad esempio, alla possibilità di installare impianti fotovoltaici nelle strutture turistiche all'aumento di 8 milioni di euro del fondo unico per lo sport, con l'obiettivo di aiutare le associazioni e le società sportive dilettantistiche, che nei territori rappresentano il cuore di chi promuove lo sport come strumento di benessere e salute. c'è il sostegno dei piccoli Comuni italiani. Altro capitolo è invece la sanità, per la quale si stanziano circa 1,1 miliardi di euro per evitare che il problema del cosiddetto *payback* sui dispositivi medici finisca per affossare le aziende del settore biomedicale. Molto positiva è la costituzione dei posti fissi di Forze dell'ordine nelle strutture ospedaliere con reparti di emergenza e urgenza, sulla base di una valutazione che verrà chiaramente effettuata dal questore competente. La cronaca ce lo ricorda. Ad esempio, a Vicenza, pochi mesi fa un'infermiera è stata aggredita e ferita al pronto soccorso dell'ospedale San Bortolo. Da troppo tempo leggiamo di aggressioni assurde e ingiustificate, che mettono a rischio l'incolumità fisica di coloro che lavorano per tutelare la salute di tutti noi. Un altro tema, sempre in ambito sanitario, è quello della carenza di personale ospedaliero nei reparti di emergenza e di urgenza.

di rimanere volontariamente in servizio. Siamo consapevoli che queste e altre soluzioni sono assolutamente temporanee, però il problema della carenza di medici, infermieri e personale sanitario è strutturale e questo Governo lo eredita, purtroppo, dal passato. Andrà affrontato con una seria programmazione, valorizzando le risorse interne, evitando le distorsioni del sistema attuale, ma sapendo che abbiamo di fronte un grande obiettivo: difendere la sanità pubblica che - lasciatemi dire è un patrimonio di tutti, perché tutela la salute di ciascuno di noi. Mi avvio alle conclusioni. A chi pone muri ideologici, ad esempio con le derive ambientaliste, lancerei oggi un messaggio: con la politica dei no questo Paese è rimasto fermo, ma col centrodestra al Governo si cambia registro. Nel sottosuolo italiano ci sono potenzialmente dieci miliardi di metri cubi di gas; su questo punto sono convinto che è doveroso dare risposte serie, non demagogiche, individuando soluzioni, definendo una strategia energetica sostenibile a 360 gradi, da un punto di vista ambientale, economico e soprattutto sociale. Il provvedimento in esame conferma il nostro approccio concreto. Il Governo ha fatto bene, questa maggioranza lo sostiene convintamente. Andiamo avanti su questa strada. Per questo motivo il Gruppo Civici

dare risposte strutturali (poi cercherò di spiegarle nel merito) alle problematiche che abbiamo, che non si risolvono dalla sera alla mattina e che - come ho detto altre volte - non sono colpa

Alla Camera avete approvato in Commissione addirittura la stabilizzazione di una parte dei ricercatori precari; avete scoperto che la misura non era coperta dal punto di vista economico e l'avete stralciata.

In sostanza non fate mai un intervento strutturale su questo terreno. Il tema degli extraprofitti serve anche perché sulla questione energetica bisogna intervenire, come rilevato stamattina da un senatore nel suo intervento,

che lo Stato vada incontro al contribuente. Ma chi va incontro ai pensionati e ai lavoratori dipendenti che pagano fino all'ultimo centesimo? Sono gli uni che in questo Paese pagano realmente le tasse! Chi gli va incontro? Questo

oltre i profitti. Non penso che l'impresa sia un soggetto che fa della beneficenza; so benissimo che ha bisogno di avere una redditività per poter investire. Siamo

un decreto così importante da aver visto anche un apporto costruttivo delle minoranze, a partire dal Gruppo cui appartengo, Italia Viva e Azione, perché, quando si parla di bollette, di carovita, di energia, del benessere delle famiglie, delle imprese e della crescita, saremo sempre dalla parte di chi vuole costruire politiche attive e propositive per il Paese. *(Applausi)*. Invece no, non abbiamo avuto questa possibilità, perché con la sono venuti meno anche gli apporti costruttivi da parte di tanti emendamenti. Prima di tutto, vorrei sottolineare quello che manca in questo decreto-legge. Ci sono due questioni, di merito e di metodo:

la situazione drammatica che stiamo vivendo. Basta andare in qualsiasi ospedale o pronto soccorso per capire quello che sta succedendo, anche nei luoghi dove la sanità funziona bene.

Avete criticato tanto il Governo Draghi, perché era un Governo dei tecnici e non c'era la politica, ma poi in realtà abbiamo visto che quel Governo ha fatto tante riforme e ha messo molti soldi proprio per le priorità del Paese. stati la crescita e soprattutto l'aiuto e il sostegno alle imprese, che sono state le prime a darsi da fare, come hanno sempre fatto, senza lamentarsi. quel Governo ha stanziato risorse importanti, quindi questo era il momento di dimostrare davvero che la politica potrebbe innalzare il livello, l'asticella, e fare qualcosa di concreto.

come sia mancato il tema della responsabilità nell'approccio a questo decreto-legge, ma non solo. Pensiamo a quello che è accaduto nei giorni scorsi con l'alluvione in Emilia-Romagna, che ha visto tante vittime, tanti sfollati e tante famiglie in difficoltà. A tale riguardo, avevamo chiesto, come Italia Viva e Azione, di ripristinare immediatamente la cabina di regia Italia Sicura. Non l'avete fatto e non ci avete ascoltato neanche di fronte ai drammatici, tragici avvenimenti che ci sono stati.

Penso in modo particolare al Fondo sui farmaci innovativi, che ha un avanzo che abbiamo chiesto anche al Governo di poter utilizzare subito, non avrebbe oneri aggiuntivi per lo Stato dato immediatamente una risposta sulla disponibilità di questi farmaci, a cominciare da quelli salvavita,

Quindi anche questa è una grande opportunità. Abbiamo dato anche la nostra disponibilità a rivedere tutta la questione legata al *payback*, ma anche in tale materia alcune questioni non sono state affrontate.

dalle parole del ministro Fitto nei giorni scorsi, che forse tutte le risorse a disposizione per il PNRR non saranno spese nei tempi utili. Quando ci capiterà di nuovo l'opportunità

il lavoro o la preoccupazione di come arrivare a fine mese e pagare le bollette. C'è poi la preoccupazione di tanti giovani, che hanno un disagio enorme, soprattutto dopo il Covid. Anche su questo abbiamo chiesto grande responsabilità, perché servono davvero politiche di aiuto e di sostegno al disagio mentale e alla preoccupazione per il futuro,

Ci auguriamo però che la prossima volta, con altri decreti importanti che sono in arrivo, si possa davvero discutere nel merito e magari anche accogliere tante proposte che vengono dalle minoranze: parlo, per quanto mi riguarda, di Azione-Italia Viva-RenewEurope.

al nostro esame - come tutti ben sanno - è entrato in vigore il 1° aprile, quindi ha già in larga parte dispiegato i propri effetti, che erano e rimangono quelli di dare un sostegno concreto alle famiglie e alle imprese più colpite da questa crisi energetica. Molte altre disposizioni sono state aggiunte ed altre sono state affinate durante l'esame della Camera, che noi abbiamo fortemente condiviso. Il risultato è un insieme di norme equilibrate che dosano le opportune risorse economiche. La *ratio* del Governo è risultata quanto mai appropriata: non si sono semplicemente replicate le norme precedenti, ma sono state cucite su misura sulle necessità del tessuto sociale italiano e sui bisogni riscontrati.

Si prosegue con misure di sostegno mirate, perché - come tutti ben sappiamo e proviamo sulla nostra pelle - le risorse sono scarse, ma nonostante questo e malgrado una manovra economica fatta solo pochi mesi fa, il decreto-legge mette in campo interventi per la rispettabile somma di circa 5 miliardi di euro. Bene quindi ha fatto l'Esecutivo a non anticipare a dicembre le misure per tutto l'anno, ma a immaginarne di nuove alla scadenza dei vecchi sostegni che terminavano a marzo e quindi più appropriati e consoni ai bisogni che si sarebbero riscontrati nell'inizio dell'annualità. Quindi, le nuove misure sono ora più puntuali e ottimizzano le risorse economiche impiegate. L'obiettivo è sostenere le famiglie, infatti è stata ora ampliata la platea di quelle che possono beneficiare della tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica. Viene confermato il *bonus* sociale per i cittadini che si trovano in una condizione di disagio economico e l'obiettivo ulteriore era ed è quello di sostenere i settori produttivi, anch'essi provati dai rincari energetici. Ebbene, come abbiamo visto dalle ultime proiezioni della Commissione europea, l'Italia cresce e cresce oltre la media europea. Per le imprese è stato prorogato il riconoscimento di alcuni crediti di imposta, ma è prevista anche la rideterminazione della base imponibile ai fini del calcolo del contributo di solidarietà temporaneo, in particolare rivolto ai soggetti che producono, importano o vendono energia elettrica, gas naturale o prodotti petroliferi. Vengono introdotte disposizioni per facilitare la produzione di agroenergie. (Ismea) potrà ora dare garanzia diretta per i finanziamenti a micro, piccole e medie imprese agricole e della pesca, che investono nell'autosufficienza energetica e nella riduzione dei costi di approvvigionamento energetico. Questa, in particolare, è una norma concepita e voluta da Forza Italia. Il decreto affronta inoltre le criticità del Servizio sanitario nazionale emerse soprattutto durante l'ultimo anno e sfida il problema delle liste d'attesa, che sono ancora troppo lunghe anche per la mancanza di medici e di infermieri.

Inoltre, viene messo in primo piano il tema dei medici che decidono di andare in pensione prima del tempo, ma il problema più grande è quello dei medici italiani che migrano, in cerca di occasioni migliori non offerte dal nostro Servizio sanitario nazionale. Andrà risolto, perché non possiamo permetterci di perdere professionalità che si sono formate da noi, costi nostri e investimenti nostri, e poi vanno all'estero (fuggono, se si può dire anche questo). Oltre a ciò, si immagina di istituire appositi presidi di polizia negli ospedali per fermare le aggressioni ai medici e agli infermieri nei pronto soccorso.

Ancora più intollerabile è che un medico donna o un'infermiera debbano avere paura di dare la propria disponibilità a svolgere un turno notturno in ospedale: anche a questo va posto rimedio. Nel decreto vengono inoltre messe in campo misure per superare il cosiddetto *payback* sui farmaci. Da ultimo, il decreto, che era strutturato in tre capitoli, affronta il campo fiscale, in cui pure sono state adottate diverse misure: vengono ridotte le sanzioni e definiti, con modalità agevolate, gli avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione e atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili al 1°gennaio 2023. Ugualmente, vengono modificati alcuni termini degli istituti deflattivi del contenzioso e di definizione agevolata, che erano stati disciplinati dall'ultima legge di bilancio. Quindi sono previste altre misure per andare incontro al contribuente e iniziare un nuovo percorso di conciliazione con il fisco; è evidente il tentativo di anticipare quello che sarà il nuovo approccio dello Stato nei confronti del contribuente, che verrà delineato dalla riforma fiscale concepita da questa maggioranza.

come al solito, con il vostro solito scaricabarile, date la colpa all'ARERA, così come in legge di bilancio, quando non avete rinnovato lo sconto sulle accise, avete dato ai benzinai la colpa dell'aumento del costo dei carburanti. Avete promesso per mesi di riscrivere il contributo sugli extraprofitti energetici e invece l'avete peggiorato, perché avete ridotto la base imponibile, tagliando il contributo e facendo perdere 400 milioni di euro. di euro. Confermate quello che abbiamo già visto in questi mesi, cioè che vi siete candidati ad essere i Robin Hood al contrario. Robin Hood infatti toglieva ai ricchi per dare ai poveri; voi invece togliete ai poveri e strizzate l'occhiolino ai ricchi. Anche in questo decreto-legge avete strizzato l'occhiolino agli evasori, inserendo uno scudo penale per omessi versamenti di IVA maggiori di 250.000 euro. Non dite che sono piccoli contribuenti: più di 250.000 euro significa un fatturato che supera il milione di euro.

del ministro Giorgetti. Che fine hanno fatto quelle dichiarazioni? Forse vi spaventano le proteste dell'associazione bancaria? Vi suggerisco di leggere le dichiarazioni dell'amministratore delegato della più grande banca italiana, Intesa San Paolo, che si dice disposto a pagare un contributo sugli extraprofitti bancari, che, secondo «Il Sole 24 Ore», nel primo trimestre 2023 sono aumentati fino al 200 per cento. Vi avevamo proposto di prendere questi extraprofitti e di creare un fondo per sostenere le famiglie nel pagare i mutui. Forse i mutui. Forse non ve ne state accorgendo, ma oggi c'è un Paese allo stremo: il numero dei poveri assoluti è il più alto di sempre (più di 5 milioni), 4 milioni e mezzo di lavoratori non riescono a uscire dalla condizione di povertà e i divari non fanno che fanno che aumentare. E voi, con questo Paese allo stremo, continuate ad accanirvi sui più deboli. Avete tolto il reddito di cittadinanza, quindi avete penalizzato i poveri; avete tagliato ai pensionati in legge di bilancio; avete tolto alle imprese due strumenti fondamentali che erano serviti a far ripartire l'economia (penso al superbonus e a Transizione 4.0). Avete tagliato anche i fondi per gli in legge di bilancio avete tagliato il fondo affitti, il fondo morosità incolpevole e il fondo affitti per gli studenti fuori sede (infatti, gli studenti oggi sono accampati nelle tende fuori dalle università e vi chiedono di rifinanziare quel fondo; e noi ve lo chiediamo con loro). di quegli affitti non volete parlare e invece parlate di affitti inesistenti, come l'affitto dell'utero, che è già un reato in questo Paese. *(Applausi)*. Vi voglio dare questa notizia: l'utero in affitto in Italia è un reato. quasi provate a farlo passare come la causa della denatalità, perché anche in questo caso non avete il coraggio di affrontare il problema. La causa della denatalità è la precarietà lavorativa; la causa della denatalità è la mancanza di servizi e di sostegno alle famiglie, che non riescono a conciliare la vita lavorativa con quella familiare, perciò non fanno figli. Passiamo alla parte sulla sanità. Anche qui siete riusciti a fare una retromarcia clamorosa, sconfessando il vostro stesso Ministro. In realtà, io apprezzo il tentativo che aveva fatto il Ministro, volto a porre un argine all'esternalizzazione verso la sanità privata e un limite all'utilizzo dei gettonisti. gettonisti. Evidentemente, però, quella parte di maggioranza che invece preme per l'esternalizzazione e per la privatizzazione della sanità, perché nelle Regioni in cui governa la sanità è tutta privata, è riuscita a far passare la sua linea. In questo momento, se non ve ne siete accorti, la sanità è la vera emergenza di questo Paese.

le Regioni a farlo. Invece anche qui, sconfessando il Ministro, avete fatto una retromarcia clamorosa, addirittura ampliando l'utilizzo dei gettonisti ad altri reparti, non solo a quello del pronto soccorso, e poi, ancora più geniale, prevedendo più contributi affinché i medici possano fare più straordinari. Allora forse non avete capito che il problema non sono gli straordinari. Il problema è la mancanza di medici, che già fanno turni massacranti, pertanto chiedere a loro di fare più straordinari è vergognoso

proprio perché manca il personale. Quindi, quelle poche risorse andrebbero investite tutte per la stabilizzazione del personale precario e per l'assunzione di tutto quel personale che in questo momento è esternalizzato e lavora presso le cooperative. Voi, però, avete deciso di non investire un euro in sanità. Lo abbiamo visto in legge di bilancio. Avevate promesso di arrivare all'8 per investito in spesa sanitaria, come gli altri Paesi europei. Noi, con fatica, in pandemia avevamo raggiunto il 7 per cento; voi, in previsione, state scendendo al 6,2 per cento nel 2025, quindi meno di quello che si investiva prima della pandemia. Infine, tutto questo lo state portando avanti mentre coltivate progetti che andranno ad approfondire le disuguaglianze alle quali accennavo prima.

vi dice di fare attenzione perché, com'è ovvio e come vi diciamo da tempo, a costo zero non si potranno garantire i livelli essenziali di prestazione su tutto il territorio nazionale. Servono 100 miliardi: questa è la stima Svimez. La Commissione europea, però, prevede anche un danno per le casse dello Stato, quando permetterete alle Regioni di trattenere il proprio gettito fiscale. Per questo, proprio per approfondire i profili finanziari dell'autonomia differenziata di tale progetto scellerato, noi oggi abbiamo chiesto un'indagine conoscitiva in Commissione bilancio. Tutto questo lo state facendo solo per aver promesso di regalare un vessillo elettorale alla Lega prima delle elezioni in Lombardia e adesso, nel silenzio compiacente di tutti gli alleati di Governo, state portando avanti questo progetto scellerato. Vorrei allora concludere con le parole che ha citato il Presidente della Repubblica evocando Manzoni in occasione dei centocinquant'anni dalla sua morte: «Ambiva a un'Italia unita, che non fosse una mera espressione geografica, una addizione a freddo di diversi Stati e staterelli, ma la sintesi alta di un unico popolo, forte e orgoglioso della sua cultura, della storia, della sua lingua, delle sue radici No, non c'è più differenza tra l'uomo delle Alpi e quello di Palermo». Nell'annunciare il voto contrario del mio Gruppo, vi vi prego di riflettere, finché siete in tempo, prima di consegnare questo Paese alla disgregazione e vi esorto a diventare davvero i patrioti che dite di essere.

questo Governo ha tentato di affrontare fin da subito, con misure concrete, che vadano davvero ad incidere per aiutare le famiglie e le imprese.

con chiarezza che questo è uno dei tanti tasselli e dei tanti interventi che in soli sette mesi il Governo ha portato alla luce. Vediamo quindi più nello specifico alcuni fra i più importanti interventi che sono previsti in questa nuova norma. Per il secondo trimestre del 2023 ci saranno agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica per i clienti domestici economicamente svantaggiati, che ARERA rideterminerà per un limite di 400 milioni di euro. Viene prorogata la riduzione dell'aliquota IVA al 5 per cento alle somministrazioni di gas metano usato per combustioni per usi civili e industriali, per i consumi nei mesi di aprile, maggio e giugno del 2023. Si prevede la riduzione del 5 per cento dell'aliquota IVA anche in relazione alle forniture di servizi di teleriscaldamento, nonché alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia. Vengono poi stanziati 280 milioni per la riduzione degli oneri generali di sistema del settore gas a carico delle utenze nel secondo trimestre dell'anno in corso. Si prevede la possibilità di erogare un contributo nei mesi da ottobre a dicembre del 2023 a parziale compensazione delle spese sostenute dalle famiglie per le spese di riscaldamento e qui

appunto per la componente energetica nel secondo trimestre del 2023; di un credito d'imposta per le imprese dotate di contatore di energia elettrica di specifica potenza disponibile diverse dalle energivore, con un contributo pari al 10 per cento; di un credito d'imposta per le imprese gasivore, anche qui in misura del 20 per cento, e di un credito d'imposta per l'acquisto di gas naturale le imprese non gasivore pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato nel secondo trimestre di quest'anno. Sono tutti interventi concreti che vanno ad alleviare un problema, che è quello del costo dell'energia per imprese e famiglie, che purtroppo in questi mesi si è ulteriormente aggravato, ma non finisce qui: si incrementa di 10 milioni di euro il fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, da destinare all'erogazione di contributi a fondo perduto per associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi e piscine per fronteggiare l'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica. elettrica. Un altro intervento molto importante è quello relativo all'articolo 5, che ridetermina la base imponibile ai fini del calcolo del contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 per i soggetti che producono, importano e distribuiscono energia elettrica e gas naturale o prodotti petroliferi, prevedendo l'esclusione dell'utilizzo di riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione di imposta o destinate alla copertura di vincoli fiscali, che siano parimenti escluse dal calcolo della media dei redditi complessivi conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al primo gennaio 2022. In un'altra disposizione introdotta alla Camera è previsto un credito d'imposta per le *startup* operanti nei settori dell'ambiente, delle energie rinnovabili e della sanità, per le spese sostenute in attività di ricerca volte a garantire la sostenibilità ambientale e la riduzione dei consumi energetici. Si tratta quindi di tante misure che vanno nella direzione - lo ripeto - di ridurre i costi per famiglie e imprese.

ancora impugnabili al primo gennaio 2023. Si tratta di una serie di semplificazioni dal punto di vista fiscale per i soggetti che sono stati oggetto di avvisi di accertamento o di avvisi di rettifica e liquidazione, che vanno ulteriormente a semplificare il rapporto tra il cittadino e il fisco. È uno dei tanti interventi ai quali seguirà, come tutti ben sanno, l'approvazione della delega fiscale, attualmente in discussione alla Camera. Camera. Nel complesso stiamo parlando di un atto normativo assolutamente necessario in un momento molto critico e molto difficile, che prevede interventi mirati e specifici che, da un lato, agevolano il rapporto il rapporto tra i cittadini e il fisco e, dall'altro, danno concretamente una mano alle nostre imprese e alle nostre famiglie, che in questi mesi hanno subito rincari energetici notevoli. In quest'ottica il Governo, che ha iniziato il proprio percorso sette mesi fa,

un conto è chiedere alle opposizioni un atteggiamento collaborativo per un andamento celere dei lavori, altra cosa è chiedere di licenziare più di cento emendamenti in pochi minuti. Questo è francamente inaccettabile e lo è ancora di più su un provvedimento nato per dare continuità agli interventi contro il caro energia, ma che alla fine si è ritrovato a intervenire su così tante materie che si fatica a comprendere la *ratio* che ne è alla base e soprattutto le strade che sono state imboccate. Pensiamo alle norme sulla sanità. Tutte le forze politiche durante la pandemia avevano elogiato i nostri operatori sanitari, tanto che per la prima volta sembrava maturata una consapevolezza trasversale sull'importanza della sanità pubblica; invece, ancora oggi si continua a non dare le risposte che il servizio sanitario attende, a partire dal rafforzamento della spesa sanitaria, con l'obiettivo di avvicinarci all'8 per cento del PIL, mentre, come sappiamo, stiamo scivolando verso il 6 E poi le assunzioni e la stabilizzazione del personale sanitario sono l'unico modo per contrastare i fenomeni di abbandono ad appannaggio delle strutture private e delle attività libero-professionali, oltre che del progressivo invecchiamento del personale medico. Questa è la strada che dovremmo intraprendere per rispondere al drammatico tema delle liste d'attesa in un Paese in cui, come ci ha detto ieri Eurispes, per colpa del carovita, un italiano su quattro ha rinunciato a fare visite e controlli. E invece, con questo provvedimento si continua a percorrere la strada delle chiamate a gettone, che ingrossa le sacche del precariato e non garantisce quella continuità nelle cure che è un requisito essenziale della qualità delle prestazioni. Un tempo si sarebbe detto che in questo modo il privato prenderà il posto del pubblico, ma qui siamo oltre, perché la sanità privata non ha interesse a investire nei piccoli centri o su prestazioni a basso margine di profitto. Questi servizi, come la medicina di base, può garantirli solo il pubblico, e per questo ci saremmo aspettati ben altri interventi, come la previsione di ulteriori risorse per il rinnovo del contratto nazionale di di lavoro per gli anni 2022-2024; l'impegno a trovare risorse per superare il blocco del *turnover*, come tra l'altro annunciato dal Ministro della salute nell'illustrazione delle sue linee programmatiche. Il provvedimento non fa meglio su altri punti. Contro il caro bollette per le famiglie si è scelto di procedere con una parziale proroga di parte delle misure in essere, senza alcun impegno alla stabilizzazione o alla programmazione. Una coperta clamorosamente corta, davanti a un aumento del costo delle bollette stimato in 300 euro a famiglia e soprattutto al fatto che - cito sempre Eurispes - il 62 della popolazione di un Paese mediamente anziano e con numerose zone climaticamente svantaggiate ha spento il riscaldamento e rinunciato all'acqua calda. C'è poi il grande tema delle imprese, per le quali, nonostante la diminuzione dei costi delle materie prime, l'aumento delle bollette per il 2023 si fissa in un +35 un aumento che incide soprattutto sulle imprese energivore e gasivore, che oggi arrancano nella competizione con le imprese di quei Paesi in cui il prezzo dell'energia è più basso. Eppure, gli spazi per recuperare le risorse c'erano, a partire dai miliardi degli extraprofitti accumulati dalle società energetiche nel 2022, incredibilmente operato per un restringimento del contributo di solidarietà da parte di questi soggetti e un'ulteriore riduzione è avvenuta proprio con questo provvedimento. È altresì doveroso sottolineare, Presidente, interventi legati al sistema fiscale: mi riferisco alla norma sulla previsione di nuove cause di non punibilità per alcuni reati tributari e a quelli sulla regolarizzazione con il pagamento di sanzioni ridotte per attività finanziarie estere e sugli immobili situati all'estero. una norma - quella sugli immobili - che ha il sapore di una beffa, perché ricorda la bocciatura dello schema del certificato europeo di filiazione, che avrebbe garantito ai figli di coppie omogenitoriali diritti ereditari omogenei su tutto il territorio europeo. Detto in altri termini, se qualcuno non ha dichiarato un immobile all'estero, può tranquillamente regolarizzarlo; se lo eredita il figlio di una coppia omogenitoriale avrà problemi a farlo, ma ancor più grave è il messaggio che viene veicolato: anziché operare per un patto virtuoso tra fisco e contribuenti, si strizza l'occhio a un modello vizioso, quello in cui lo Stato tollera o addirittura offre copertura al mancato rispetto delle regole, con buona pace di tutti i contribuenti onesti. Come se non bastasse, il Governo ha anche ritirato le misure contro il caro affitti per gli studenti universitari, su cui in questi giorni è stato un profluvio di dichiarazioni tra il paternalistico e l'insofferente, senza capire che il problema di uno studente è prima di tutto il problema di una famiglia; anzi, è la principale preoccupazione Insomma, Presidente, dove sono in questo provvedimento le tanto celebrate famiglie? Dove sono le risposte ai tanti interrogativi che si pongono nelle case degli italiani (il carovita, la possibilità di vedere i propri figli studiare o l'idea di avere alle spalle un servizio sanitario adeguato)? Questo provvedimento risponde poco e male; in alcuni casi, riesce addirittura a peggiorare la situazione, alimentando un clima di incertezza, se non di diffidenza, verso lo Stato e le sue articolazioni. Ancora una volta, al di là dei proclami, questo Governo dimostra di non avere una programmazione o una visione per rispondere alle preoccupazioni degli italiani. Per questo motivo, Presidente, annuncio il voto contrario del Partito Democratico.

ma auspichiamo che il Governo tenga conto del suo contenuto. Se sarà necessario, potremo comunque ripresentarlo nell'ambito di un altro provvedimento, perché ci sta particolarmente a cuore.

perché avete parlato di tutt'altro, ma poco del decreto-legge n. 34 del 2023. Il provvedimento mette in campo 4,9 miliardi di euro: per alcuni non sono tanti, ma in questa situazione di gravità sono tantissimi. Vorrei fare un parallelo: ognuno di noi in quest'Aula ha partecipato a delle competizioni elettorali per il rinnovo dei consigli comunali. Mi riferisco ai piccoli Comuni, dove un sindaco viene eletto, governa per cinque anni se ha governato bene, nella maggior parte dei casi viene riconfermato; ma, se ha governato male - banalmente, se non ha coperto tutte le buche presenti sulle strade - viene battuto dal suo avversario.

Voglio dire che in 72 sedute del Senato avete raccontato di un Paese che è in catalessi e avete fatto bene, perché è vero, avete ragione: il nostro Paese è

ancora le imprese energivore; inoltre, per esempio per la mia Sardegna e per la Sicilia istituisce un fondo di aiuti alle imprese particolarmente energivore che, se ce ne sarà bisogno, andrà sicuramente rimpinguato.

questioni sanitarie, la riforma ci sarà. Il Governo Meloni governerà per cinque anni e farà una reale riforma del Sistema sanitario italiano. Farà non interventi *spot*, ma riforme vere. Noi abbiamo un'eredità pesante, cara Presidente: abbiamo una mancanza di medici che qualcuno oggi ha stimato in 300.000 unità unità e una carenza di personale sanitario ancora più elevata. Vorrei ricordarvi alcuni numeri: dal 2001 al 2023 su 13 Ministri dell'università, tre sono imputabili al centrodestra; dal 2001 al 2023 quattro Ministri su 11 sono imputabili al centrodestra, tutto il resto è del centrosinistra. Ciò significa che quello che abbiamo ereditato sulla sanità è dovuto al fatto che voi non avete avuto una minima visione. La collega Lorenzin, ministro della sanità, è stato il Ministro con il mandato più duraturo: avrebbe potuto stravolgere in meglio la sanità italiana, ma ciò non è accaduto. Siamo nella situazione che voi avete raccontato, cioè in un totale disastro. Non dovevate prevedere la pandemia, ne avreste potuto banalmente aggiornare in maniera elastica il numero di laureati in medicina e di specializzandi, prendendo due dati: il numero di pensionamenti a venire e lo spopolamento dalle zone interne verso le città. Ad esempio, se avessimo rimodulato l'attività e il reclutamento dei medici di base, non ci troveremmo in paesi come il mio, un paese collinare della Sardegna, in cui mancano i medici di base ormai

Quindi ben vengano, ancora e purtroppo, i medici gettonisti e l'incremento della tariffa oraria per chi fa gli straordinari. Ricordo infatti che, se un medico vuole fare lo straordinario, è giusto che venga ben pagato. Poi ci sono i medici che lo straordinario non lo vogliono fare e va bene lo stesso. Chi però fa lo straordinario deve essere ben pagato. Ben vengano il riconoscimento dei titoli professionali conseguiti all'estero, il contrasto agli episodi di violenza nei confronti del personale sanitario, la deroga alla compatibilità per il personale delle professioni infermieristiche: qualcosa che stavamo attendendo da tempo. Vorrei ora parlare di *payback*. Su 4,9 miliardi, stati messi un miliardo e 85 milioni *payback*. Ho sentito, da parte non di tutti i colleghi, che era corretto mettere un aiuto su questo provvedimento che probabilmente andrà ad ammazzare svariate centinaia di piccole e medie imprese. Il *payback* nel 2015 con il ministro Lorenzin, il ministro Padoan all'economia e con il Governo Renzi lo avete votato voi. aiuti del 2022 avete messo voi l'attivazione del *payback*, non l'abbiamo messa noi. Vorrei semplicemente ricordarvelo. Quindi, oltre a migliorare il decreto-legge aiuti sul caro energia, lo miglioriamo anche sul *payback*. Lo avete attivato e noi cerchiamo di disinnescare una bomba a orologeria e non solo per le piccole e medie imprese, ma anche per le nostre strutture sanitarie.

in cui verrà attivato il MES; la politica italiana dovrebbe mettersi al fianco del presidente Meloni e chiedere in questo momento una riforma di quello strumento, invece di attaccare sempre e comunque il fatto che noi non abbiamo ancora dichiarato che lo andiamo a sottoscrivere. Tutto ciò avendo visione chiara al fianco degli italiani e non contro gli italiani, come avete fatto voi, riducendo l'Italia allo stato in cui è. Quando raccontate che l'Italia è in questo stato, vuol dire che avete lavorato

Si pensa alle vittime dell'amianto. Ricordo che il Governo Conte aveva dato alle Regioni dei milioni di euro per togliere l'amianto, ma non dava neanche un centesimo alle Regioni

Questo è uno sbaglio che fate perché non amministrate mai una Regione e un Comune; e dove lo fate, magari venite commissariati, come accade spesso. Il "metodo Giuseppi"... visti gli interventi di ieri, è per non costruire: non volete costruire il ponte che collega la Calabria e la Sicilia e non volevate ricostruire le scuole italiane, a cui chiedevate di togliere i tetti. Voi siete contro l'evoluzione. State tranquilli perché, se ci fosse stato il ministro Salvini, il risarcimento ci sarebbe stato comunque. Alla collega Castellone, per il suo tramite, signor Presidente, vorrei dire solo una cosa sullo sconto delle accise. In pochi mesi abbiamo dimostrato di avere ragione.

E mi fa piacere se, grazie all'intervento della collega Castellone, oggi abbiamo dimostrato che chi ci ha preceduto non ha abolito la povertà. *(Applausi)*. Dichiaro il voto favorevole di Fratelli d'Italia sul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

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza. Estraggo ora a sorte

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'articolo unico del disegno di legge n. 714, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34,

Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge

al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Nel marzo 2017 è stato firmato l'Accordo quadro tra Italia e Canada sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione, indispensabile per poter concludere gli accordi di dettaglio con le singole Province e i territori canadesi. A pochi mesi di distanza dalla firma dell'Accordo quadro tra i due Stati, sono iniziati i contatti tra il Governo della nostra Repubblica e quello della Provincia del Québec, volti a definire un primo protocollo d'intesa fortemente - ripeto, fortemente - auspicato sia dai cittadini italiani residenti in quella Provincia (un numero che aumenta ogni anno), che dai cittadini quebecchesi residenti in Italia. L'*iter* procedurale per la definizione dell'intesa tecnica tra Italia e Québec per la conversione delle patenti è da oltre sei anni allo studio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in collaborazione, come già detto, con il Ministero degli affari esteri Nel 2021 la Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha ulteriormente formalizzato le richieste di chiarimenti da presentare alle autorità quebecchesi, per il tramite del MAECI; chiarimenti necessari per la prosecuzione dei negoziati. Sostanzialmente, dopo sei anni dall'inizio dei negoziati e nonostante i diversi contatti intercorsi tra le autorità delle due parti, nonché le mie sollecitazioni avanzate a livello parlamentare, non si è finora pervenuti ad alcuna conclusione, né risultano prospettate ipotesi temporali relative alla conclusione delle trattative. Nell'interrogazione presentata oltre quattro mesi fa, chiedevo ai Ministri in questione se avessero ricevuto dalle autorità quebecchesi riscontri relativi alla prosecuzione dei negoziati, quali siano gli ostacoli tecnici che ancora impediscono di arrivare alla conclusione dell'*iter* ed entro quanto tempo ritengano di poter chiudere il protocollo d'intesa, la cui prolungata conclusione conclusione sta suscitando notevoli disagi ad una platea sempre più larga di cittadini. A queste mie domande non ho mai ricevuto risposta, nonostante sappia per certo che i tecnici del Ministero abbiano fornito tutte le informazioni necessarie ai diretti interessati per rispondere alle mie richieste. Tutto tace, come si suol dire, eppure credo che il nostro lavoro di parlamentari sia quello di cercare di dare soluzioni strutturali ai cittadini, in Italia come all'estero. Auspico quindi una pronta risposta alle mie domande, ma soprattutto a quelle dei cittadini, che attendono da anni un cenno dalle istituzioni.

per la dolorosa dipartita di un nostro concittadino che nel cuore della notte si è tolto la vita lanciandosi dal quarto piano della propria abitazione. Alla base del gesto, la perdita del posto di lavoro, che ha gettato l'uomo in uno stato di sconforto e lo ha condotto ad aprire la finestra del suo balcone. Vada alla famiglia il mio più sentito cordoglio. Onorevoli colleghi, la perdita del lavoro è un evento traumatico e doloroso che può avere ripercussioni devastanti sulla salute psicofisica delle persone, potendo rappresentare una sconfitta, un fallimento, una rottura nel tessuto delle relazioni sociali e familiari. Già nel 2012, secondo il rapporto Osservasalute, si registrava un incremento dell'utilizzo degli psicofarmaci, come effetto del disagio scatenato dalla difficoltà socioeconomica e un aumento dei suicidi per la perdita del lavoro, rispetto al passato. A distanza di anni, purtroppo, il *trend* è aumentato ancora di più, e ormai la perdita occupazionale va considerata come una causa diretta di suicidi. suicidi. Noi, istituzioni, non possiamo restare inerti di fronte a questa tragedia che, negli ultimi dieci anni, ha spinto oltre 1.000 italiani a togliersi la vita per motivi economici. Abbiamo il dovere civico e morale di levare la corda di mano a chi non è riuscito a sostenere tutto il peso e la vessazione di un sistema economico e lavorativo che sta rendendo i ricchi sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri. Addirittura, nel Mezzogiorno, i casi di suicidio sono balzati dal 14 per cento del 2012 al 32 per cento, un incremento figlio della povertà dilagante che serpeggia in un territorio che, dal 2002 al 2017, ha spinto oltre due milioni di cittadini ad abbandonare la propria terra, più della metà giovani, di cui il 33 per cento laureati. Onorevoli colleghi, non possiamo più permettere che le persone si sentano abbandonate e senza speranza a causa della disoccupazione. Non possiamo più accettare che la mancanza di lavoro diventi una condanna a morte. Ricordiamo che la vita è preziosa e che ogni persona ha il diritto di vivere con dignità e di realizzare i propri sogni. Non lasciamo che la disoccupazione ci rubi questo diritto. Lavoriamo tutti insieme per creare una società più giusta, solidale e umana.

L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata (cosiddetto *question time*), ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento, alle quali risponderanno il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

sulle carceri del siracusano, incluso quella di Augusta, il 1° febbraio. In quell'occasione avevamo posto all'attenzione il tema rilevantissimo del sovraffollamento - da un lato - dall'altro - anche il tema del disagio psicologico, del *deficit* di sostegno sanitario e di cura psicologica in particolare, una situazione di malessere diffuso che riguardava sia i i detenuti sia il personale della Polizia penitenziaria. In quell'occasione ebbi a dire al Sottosegretario di dichiararmi parzialmente soddisfatto per la parte che riguardava gli impegni del Governo sul lato delle nuove assunzioni, dello sblocco delle assunzioni e anche di un'attenzione maggiore sulla turnazione. Mi dichiaravo però insoddisfatto sulla parte che riguardava l'attenzione da dedicare a un momento particolare e grave, che non inizia con questo Governo, perché ha riguardato già il 2022, con un *record* di suicidi (oltre 80 suicidi) che pone l'Italia al decimo posto fra i Paesi del Consiglio d'Europa. Questo è strano perché non siamo un Paese ai primi posti per i suicidi in generale, ma stiamo avanzando nelle graduatorie per i suicidi nell'ambito delle carceri. C'è un problema di fondo che va affrontato, ma mentre ne discutevamo è accaduto un altro fatto tragico. Da qui la seconda e odierna interrogazione: due persone sono decedute per sciopero della fame nel carcere di Augusta, a distanza di sessanta e quarantuno giorni rispettivamente, e una terza persona - questo l'abbiamo appreso da notizie di stampa e da quanto ha detto il Garante dei detenuti ha tentato il suicidio con impiccagione. Non abbiamo avuto notizie, il Garante dei detenuti non ha avuto notizie e neanche l'ufficio di garanzia per i detenuti ha avuto notizie di ciò che è accaduto a quelle persone. Quindi, in primo luogo vogliamo avere notizie sulla procedura, su cosa è accaduto in merito a queste vicende e, più in generale, come si intende affrontare quella che ormai è un'epidemia dei suicidi nelle carceri, che riguarda tantissime persone

senatore interrogante. Come ho già avuto modo di dire precedentemente, ogni suicidio in carcere è un fardello di dolore ineliminabile, non solo per noi del Ministero, ma per tutti noi, per la nostra coscienza e la nostra visione etica. Con riguardo ai due detenuti deceduti in ospedale in conseguenza del deterioramento delle loro condizioni, dovute presumibilmente allo sciopero della fame, sono in corso le doverose attività ispettive finalizzate all'esatta verifica di quanto è occorso nel periodo di detenzione e fino al momento del ricovero in nosocomio. Per quanto posso riferire ora, non sono emersi dei *deficit* nei doveri cui è tenuta l'amministrazione penitenziaria. Il discorso è più complesso, perché coinvolge una pluralità di competenze. Come sapete, è l'autorità regionale ad essere preposta all'assistenza sanitaria, una volta che questa non è più efficacemente erogabile all'interno del carcere. In particolare, nei limiti temporali consentiti in questa sede, riferisco che il signor Z.L.D., il primo di questa dolorosa lista, ha iniziato lo sciopero della fame il 27 febbraio 2023, ritenendo di essere detenuto ingiustamente. Il successivo 24 aprile è stato ricoverato presso l'ospedale di Augusta, ove poi è avvenuto il decesso. Dagli atti emergono delle problematiche di natura psichiatrica, tanto che, con provvedimento del 6 aprile 2023, il magistrato di sorveglianza di Siracusa aveva richiesto una precipua osservazione il successivo 17 aprile ne era stato disposto il trasferimento temporaneo presso il carcere di Barcellona Pozzo di Gotto, perché dotato di una articolazione di tutela della salute mentale. Si era in attesa del posto letto. detenuto, che chiameremo P.D., aveva intrapreso la protesta dello sciopero della fame dal 26 marzo 2023, per motivi di giustizia legati alla sua procedura di estradizione. Il 2 maggio era stato ricoverato presso l'ospedale di Siracusa, ove poi decedeva il successivo 9 maggio. È un intervallo molto breve e, quindi, sono in corso anche qui degli accertamenti per capire quali siano state realmente le cause del decesso. decesso. Siamo disposti a riferire e lo faremo sicuramente in un momento successivo, quando avremo tutta la documentazione che sta per essere acquisita.

non è un'attività obbligatoria. Non è prevista la comunicazione dell'andamento delle centinaia di manifestazioni di protesta che quotidianamente i detenuti pongono in essere sul territorio nazionale, molte delle quali cessano entro breve termine. Purtroppo è un'attività che sarebbe quasi impossibile monitorare, visto che inizia e finisce in termini spesso molto brevi. Però vi annuncio - questo è un punto d'onore - che, allo scopo di ovviare a questa problematicità, a breve sarà operativa una *mailing list* presso la sala situazioni del DAP, così che anche l'ufficio del Garante nazionale sia tempestivamente reso edotto, pressoché in tempo reale, dei fatti di particolare rilevanza che si verificheranno all'interno degli istituti penitenziari. Quindi, avremo contezza di tutti gli eventi critici, così da agevolare il miglior adempimento del proprio mandato costituzionale. Infine, per quanto riguarda la tematica dei suicidi, ribadisco l'attenzione alla sanità penitenziaria, che è e sarà massima, non nascondendo però - lo ripeto - la complessità della problematica, perché la titolarità in capo alle Regioni della competenza a organizzare ed erogare concreti servizi può creare e spesso crea un concorso di competenze. Per quanto è possibile, mi associo alla dolorosa esperienza dei familiari della persona in questione. Ripeto che, ogni volta che una persona decede in carcere, è per noi un fardello di dolore.

persone che sono private della libertà, c'è un doppio dovere da parte dello Stato stesso: quello di difendere tutti gli altri e quello di difendere innanzitutto questi cittadini, perché una sconfitta lì è una sconfitta della democrazia e di ciascuno di noi. Nello stesso tempo, pur conoscendo la sua sensibilità sul tema, non posso ritenermi soddisfatto, per un motivo molto semplice, anzi per due motivi. Il primo è che ho visitato quelle carceri il 24 dicembre e ho presentato un'interrogazione, proprio perché la ritenevo un'urgenza. La seconda è che vi sono state ripetute visite di esponenti del Governo, in particolare del sottosegretario Delmastro Delle Vedove, nelle carceri di quella zona, ma evidentemente non si è sentita l'urgenza di interventi. Questo è un tema molto delicato, sul quale evidentemente c'è un interesse che va al di là del Governo dell'opposizione. Ma quando, in alcuni casi, se n'è fatta occasione di strumentalizzazione politica, le notizie di ciò o le presunte notizie di ciò che avviene nelle carceri sono diventate oggetto anche di propaganda politica. Invece, io vorrei il contrario. Vorrei che le notizie delle emergenze, della cura di dette persone fossero qualcosa di condiviso e permettessero a tutti noi, compreso il Garante dei detenuti, di intervenire per tempo per evitare le loro morti.

Signor Ministro, nel corso della XII legislatura, la legge 103 ha delegato il Governo a procedere alla riforma delle intercettazioni. Tra i principi e i criteri direttivi cui il Governo doveva attenersi nell'esercizio della delega spiccavano quelli volti a garantire la riservatezza delle comunicazioni e conversazioni telefoniche telematiche oggetto di intercettazione, così come previsto nell'articolo 15 della Costituzione. In attuazione della suddetta delega è stato emanato il decreto legislativo n. 216 del 2017, che ha introdotto diverse disposizioni, soprattutto con riferimento alla fase della esecuzione delle intercettazioni, nonché a quella in cui i risultati delle captazioni devono essere riversati agli atti del procedimento. Anche la fase della selezione dei colloqui rilevanti è stato oggetto di specifica disciplina, in base alla quale le intercettazioni ritenute non rilevanti sono sottoposte al divieto di pubblicazione anche parziale del loro contenuto e delle stesse non può essere autorizzata la copia nemmeno se richiesto dai difensori. Nonostante questo, accade spesso purtroppo che le intercettazioni giudiziarie finiscano sulla stampa, anche quelle giuridicamente rilevanti, anche quelle fra persone non imputate né indagate. La pubblicazione delle stesse, oltre a violare il diritto di *privacy* e riservatezza, soprattutto quando le stesse concernano soggetti estranei alle investigazioni, viola anche la segretezza delle indagini in corso, a volte irrimediabilmente minate da una precoce e illegittima fuga di notizie. Considerato che si ritiene importante assicurare in maniera compiuta la riservatezza delle conversazioni e comunicazioni oggetto di intercettazioni, si chiede di sapere quali iniziative il Ministro abbia adottato abbia adottato o intenda adottare per monitorare e vigilare sulla corretta applicazione della normativa che ha riformato la disciplina delle intercettazioni e se il Governo intende intervenire al fine precipuo di garantire una maggiore riservatezza dei colloqui captati nel rispetto dell'articolo 15 della Costituzione.

sin dal primo giorno sul programma di riforme della giustizia, la disciplina delle intercettazioni, astrattamente, nel codice di procedura penale e anche dopo la riforma che l'interrogante

in un più ampio programma di revisione totale del codice di procedura penale, che noi auspichiamo essere ispirato al sistema accusatorio. Ripeto ancora una volta che noi abbiamo un codice di procedura penale, voluto da una medaglia d'argento della Resistenza, il professor Vassalli, che gode di pessima salute, in quanto demolito varie volte da interventi legislativi e dalla Corte costituzionale, anche riguardo alle intercettazioni. Paradossalmente, abbiamo un codice penale, che è ancora quello firmato da Benito Mussolini e da Vittorio Emanuele III, che gode di ottima salute e che è stato sempre ritenuto compatibile con la nostra Costituzione, benché nata dalla Resistenza. È uno dei tanti paradossi del nostro sistema giudiziario, che è completamente sfasciato.

*privacy.* In un tempo successivo, in una prospettiva più ampia di riforma del codice di procedura penale, si procederà a una radicale - e sottolineo radicale - revisione del sistema delle intercettazioni che tuteli non soltanto la *privacy*, ma anche la correttezza delle indagini e scongiuri la strumentalizzazione che spesso viene fatta attraverso la diffusione pilotata di notizie che dovrebbero restare segrete.

*(Misto-AVS)*. Signor Ministro, parto dall'articolo 5 del decreto bollette appena convertito in legge, che modifica la modalità di calcolo del contributo di solidarietà sugli extraprofitti imposto alle aziende del settore energetico, riservando loro un trattamento di favore rispetto a quello già previsto, già molto generoso; una misura che determinerà per il bilancio statale, per il solo 2023, un mancato gettito del 15,8 per cento, con conseguente relativo aggravio di oneri pari a 404 milioni. milioni. Ancora una volta, quindi, questo Governo decide di affrontare la complicatissima situazione di crisi vissuta dal nostro Paese e derivante dall'effetto della guerra in Ucraina e dalle sanzioni economiche internazionali intervenendo sugli extraprofitti con una misura redistributiva totalmente inadeguata, che dimostra asservimento ai colossi energetici del settore fossile, attingendo solo in minima parte al totale di 40 miliardi di extraprofitti accumulati negli ultimi anni. Si rinuncia quindi a incamerare somme che avrebbero potuto essere destinate a politiche energetiche diverse di transizione energetica, *in primis* quelle da investimento in fonti rinnovabili e superamento della dipendenza da fonti fossili. E non solo: gli ultimi dati ci dicono che le famiglie italiane in difficoltà economica sono più che raddoppiate rispetto all'inizio del 2022, passando dal 10 per cento dello scorso anno al 23 per cento di quest'anno. Un italiano su tre è in una situazione economica difficile, ha grosse difficoltà a pagare le bollette, uno su tre ha dovuto rinunciare alle spese mediche e all'acquisto di carne e pesce. La causa la conosciamo tutti. Siamo davanti a un'inflazione strutturale come non si vedeva da trent'anni: aumento dei prezzi, salari bloccati da decenni, precariato generalizzato. All'impennata dell'inflazione corrisponde il crollo del potere d'acquisto delle famiglie e delle persone in genere e, mentre le persone sono obbligate a pagare bollette astronomiche, le società energetiche stanno facendo grandi guadagni non previsti, anzi grandissimi guadagni che questo Governo decide di non intaccare, se non in minima parte. Ma la punta dell'*iceberg* è che, a fronte di una situazione come questa, la ricetta del Governo sembra essere acqua fresca non parlo solo degli extraprofitti: si è fatto un gran parlare delle misure sul cuneo fiscale per poi scoprire che il tutto si risolve con una *una tantum* di 500 euro che non ha continuità almeno nel 2024.

A questo si aggiunge che il lavoro atipico - ovvero tutte le forme di contratto diverso dal contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o a tempo pieno - rappresenta l'83 per cento delle nuove attivazioni, con un aumento del 34 per cento negli ultimi anni. Queste ricette ci sembrano del tutto inadeguate. Chiediamo dunque di aumentare il contributo di solidarietà sugli extraprofitti realizzati da parte delle società energetiche per destinare il relativo maggiore gettito a politiche energetiche che sostengano realmente le persone, le famiglie e le imprese italiane. oltre a queste, quali nuove iniziative intenda mettere in campo il Governo per combattere la crisi economica in atto. PRESIDENTE. Il ministro dell'economia e delle finanze, onorevole Giorgetti, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata,

facciano riferimento al contributo di solidarietà straordinario sotto forma di prelievo temporaneo per l'anno 2023, di cui alla legge di bilancio 2023, chiedono che sia aumentata sino al 100 per cento l'aliquota del contributo straordinario contro i rincari energetici di cui all'articolo 37 del decreto-legge n. 21 del 2022, che fa invece riferimento a un esercizio finanziario oggetto di bilanci già approvati. Tanto premesso, il Governo con riferimento al contributo relativo all'esercizio 2022 - è intervenuto a più riprese e, dopo un attento bilanciamento degli interessi costituzionalmente tutelati, ha fissato l'aliquota al 37 Con riferimento, invece, al contributo relativo all'anno 2023, avente una base imponibile differente, ha ritenuto di poter fissare la relativa aliquota al 50 Tale percentuale è stata oggetto di una valutazione del Governo in ordine al necessario contemperamento dei principi costituzionalmente tutelati - quali la capacità contributiva e la libera iniziativa economica - con l'esigenza di reperire tempestivamente risorse da destinare alla tutela delle fasce più deboli della popolazione. Vorrei assicurare al senatore Magni che l'attenzione continua a essere massima da parte del Governo e a breve avrà anche - credo - sorprese positive per quanto riguarda i suoi interessi. come già annunciato in sede di audizione parlamentare, alla quale il senatore Magni ha partecipato - l'intervento da parte del Governo nei confronti dei lavoratori dipendenti si è sostanziato non nei miseri 15 euro tanto declamati dall'opposizione, ma in realtà in cifre ben più consistenti, come dimostrato da da ricerche documentate anche da parte dei *media*. Concludo dicendo che prudenzialmente il Governo ha stimato l'imposta sui maxiprofitti energici, concepita da questo Governo nella legge di bilancio. Credo che a breve, quando saranno eseguiti i versamenti, avremo delle sorprese positive di maggior gettito da mettere a disposizione delle famiglie più vulnerabili.

e non hanno un extragettito, per cui riducono la loro capacità a causa dell'inflazione - perché l'inflazione c'è - e quindi perdono potere d'acquisto. Essi non sono pertanto in grado di sopperire a esigenze dal punto di vista sociale e intaccano i propri risparmi di fronte al fatto che ci sono persone che guadagnano oltre

*(M5S)*. Signor Ministro, introduco il quesito partendo da un caso particolare per giungere anche alla richiesta più ampia in relazione al potere di controllo del MEF sull'operato di Agenzia delle entrate. Si tratta del tormentato *iter* di un concorso pubblico bandito dall'Agenzia delle entrate nel 2010 per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia. Il bando è passato prima dalla dichiarazione di illegittimità, perché valorizzava tra i titoli valutabili anche gli incarichi dirigenziali a tempo determinato tramite assegnazione diretta (quindi senza concorso), di cui all'articolo 8, comma 24, del decreto-legge n. 16 del 2012, che nel frattempo la Corte costituzionale aveva dichiarato incostituzionale. Il bando poi riprendeva il suo *iter* e nel 2016 la commissione esaminatrice definiva i criteri di valutazione dei titoli; nel 2021 la graduatoria finale dell'Agenzia delle entrate veniva approvata, ma successivamente impugnata davanti al che accoglieva i ricorsi per la mancanza di un equilibrato bilanciamento nell'attribuzione del punteggio per titoli e per colloquio, come viceversa era previsto nel bando. La commissione, infatti, aveva attribuito ai titoli una valenza talmente bassa che, nell'ambito della valutazione complessiva, il loro peso risultava del tutto irrilevante, mentre la prova orale, caratterizzata da un'ampia discrezionalità valutativa, assumeva un peso determinante. Nel 2022 il TAR annullava la graduatoria. Risparmio considerazioni in merito all'obiettivo che si voleva raggiungere con questa tipologia di criteri, ma osservo che la frequenza delle impugnazioni delle procedure concorsuali, anche presso l'Agenzia delle entrate, è causa di danni alla pubblica amministrazione che, oltre a dover sopportare il costo dei giudizi, finisce per dover calibrare l'esito delle procedure selettive tenendo conto delle pronunce giurisdizionali, anche di tipo cautelare, del giudice amministrativo, a cui si aggiungono poi i ritardi nelle assunzioni e le incertezze che l'eventuale riforma della graduatoria potrebbe comportare sino allo spirare del termine per le impugnazioni. quindi quali iniziative questo Ministero ritenga di intraprendere con l'Agenzia delle entrate per evitare il ripetersi di tali circostanze; quali siano le conseguenze sull'Agenzia delle entrate a seguito dell'annullamento di una graduatoria e quali iniziative si ritenga di intraprendere per garantire la prosecuzione dell'ordinaria attività degli uffici. Chiaramente si ritiene che le procedure e le regole di reclutamento dei dipendenti pubblici dovrebbero invece garantire efficacia, trasparenza e tempi certi.

il concorso pubblico per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia fu avviato dall'Agenzia delle entrate sulla base dell'articolo 1, comma 530, della legge finanziaria 2007. La citata normativa, al fine di potenziare l'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, consentiva di procedere ad assunzioni di dirigenti per l'Agenzia delle entrate con modalità speciali di reclutamento. Tali modalità speciali consistevano, in particolare, in una deroga alla disciplina ordinaria dei concorsi pubblici per dirigente, che prevedono la valutazione dei titoli, delle prove scritte e della prova orale. Infatti, nella procedura selettiva per i 175 dirigenti oggetto della precedente interrogazione sono stati valutati i titoli previsti dal bando ed è stata espletata la sola prova orale per accertare le competenze specifiche possedute dai candidati. La procedura concorsuale è stata avviata nel 2010

Infatti il TAR del Lazio, con alcune sentenze del novembre 2022, ha parzialmente accolto i ricorsi proposti da candidati che hanno lamentato presunte illegittimità relative alla fase di valutazione dei titoli, annullando gli esiti della procedura nella parte relativa all'attribuzione del punteggio per titoli. Con il supporto dell'Avvocatura generale dello Stato è stato proposto ricorso in appello verso le predette sentenze, con istanza di sospensione degli effetti delle stesse in sede cautelare, al fine di ottenere una pronuncia definitiva sul tema nei confronti di tutti i concorrenti (vincitori, idonei e non idonei). Il 15 febbraio ha emesso le ordinanze nn. 624 e 626 del 2023, con le quali ha accolto la richiesta di sospensione delle impugnate sentenze, ritenendo che, nelle more della definizione del merito, si palesi l'esigenza di mantenere ferma la graduatoria concorsuale e fissando l'udienza pubblica per entrambi i giudizi al 16 maggio 2023. In pari data la causa è stata trattenuta in decisione e si è in attesa della sentenza alla quale l'Agenzia delle entrate si conformerà senza indugio, per assicurare la continuità dell'azione amministrativa degli uffici che ad oggi non ha registrato impatti negativi sulla prosecuzione della propria attività ordinaria. Con riferimento, infine, alla richiesta dei senatori interroganti volta a conoscere quali iniziative l'Agenzia intenda intraprendere per evitare il ripetersi di simili si rappresenta che nel 2019 sono stati pubblicati due nuovi bandi di concorso per dirigenti: 10 posti per gli uffici preposti all'attività catastale e 150 posti per gli uffici preposti alle attività di controllo e gestione dei tributi. Con l'espletamento di questi due concorsi sarà completato il reclutamento dei dirigenti che occorrono per il presidio di tutti gli uffici. Da ultimo, come indicato nel piano integrato di attività e organizzazione 2023-2025, Sezione amministrazione trasparente, l'Agenzia ha precisato che, con le vacanze derivanti dai futuri pensionamenti, intende espletare con periodicità regolare concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica dirigenziale di seconda fascia. PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica la senatrice Sironi,

in quanto il fatto di aver bandito due successivi altri bandi non risolve la questione relativa al bando precedente. La mia domanda era orientata a comprendere quali poteri di controllo e di azione possa intraprendere il MEF per garantire e controllare il corretto operato dell'Agenzia delle entrate, che evidentemente non si è comportata del tutto correttamente. Mi riterrò pienamente soddisfatta quando finalmente potrò vedere direttamente la correttezza dello svolgimento dei concorsi pubblici senza dover tutte le volte ricorrere da un tribunale all'altro. Il fatto solo che questo concorso sia durato dieci anni rileva evidentemente che qualcosa non è andato per la strada per la quale doveva andare. Tra l'altro, collegandomi anche agli obiettivi del PNRR in merito al rafforzamento dei processi di selezione

quelli che hanno più o meno la mia età ben ricordano in gioventù, ma per trenta anni ci siamo quasi dimenticati della sua esistenza. Adesso, soprattutto a seguito dei movimenti dei prezzi delle materie prime, si è assistito a un aumento dell'inflazione che non si registrava da circa trenta anni. che la causa sia soprattutto da ricercarsi sul movimento dei prezzi delle materie prime è testimoniato da autorevoli studi; l'ultimo è uscito ieri ed è di un economista considerato fra i migliori al mondo, Blanchard. Il problema è che la Banca centrale europea ha deciso da tempo di reagire a questo aumento dei prezzi con un vecchio vale a dire l'aumento dei tassi di interesse. Tale aumento, che era lo strumento da libro di testo negli anni Novanta per raffreddare un'economia che andava in surriscaldamento perché andava troppo bene e quindi portava a un aumento dei prezzi, la cosiddetta inflazione della domanda, viene applicato

al problema. Vorremmo sapere però quali sono le azioni che il Ministro intende porre in essere nelle sedi opportune per proseguire nell'azione di tutela di famiglie e imprese

reintroducendo la facoltà di rinegoziare a determinate condizioni i mutui ipotecari a tasso variabile, trasformandoli in mutui a tasso fisso e prorogando le agevolazioni fiscali e le garanzie sulla prima casa per gli *under* 36. misure hanno registrato un grande successo e dobbiamo porci anche il tema di come rifinanziarle, perché sono in via di esaurimento i relativi fondi. Per quanto riguarda l'andamento dell'inflazione e i suoi riflessi sul mercato immobiliare, a questo proposito

il riflesso sul tasso d'interesse medio sulle consistenze dei mutui delle famiglie, nella media di marzo i tassi di interesse sui nuovi prestiti per l'acquisto di abitazioni risultano pari al 4

aumenti in questo periodo. Naturalmente il Governo resta vigile sull'impatto che le condizioni di finanziamento restrittive stanno avendo e possono produrre sul mercato delle abitazioni e sul risparmio delle famiglie. Secondo gli ultimi dati disponibili, a fronte di un calo dei mutui ipotecari del 12,8 per cento nel quarto trimestre del 2022, rispetto allo stesso periodo del 2021, le compravendite di unità immobiliari a uso abitativo si sono ridotte solamente del 2,1 per cento. Questo vuol dire che evidentemente si ricorre meno all'indebitamento. Anche la dinamica dei prezzi delle abitazioni, in leggera riduzione, non mostra segnali di grande preoccupazione. Al di là delle grandezze macroeconomiche illustrate, la questione abitativa assume un particolare rilievo sociale, è all'attenzione del Governo ed è una caratteristica molto peculiare italiana. Vorrei ricordare che, nella relazione al Parlamento da ultimo approvata dalle Camere, il Governo ha destinato i margini di bilancio disponibili per finanziare, per l'anno in corso, un nuovo taglio dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti, per sopperire al fenomeno del calo del potere d'acquisto delle famiglie, in particolare quelle di reddito medio-basso. Per quanto riguarda la manovra di bilancio per il prossimo anno, che sarà oggetto della sessione di programmazione, ci sarà un'attenta valutazione considerando i dati più aggiornati sull'inflazione e sui tassi di interesse, auspicando che evidentemente con l'estate cessino gli aumenti - e ragionevolmente questo dovrebbe accadere - al fine di tutelare l'andamento del potere d'acquisto delle famiglie, del mercato del credito e l'accesso ai mutui. Il Governo - su questo concludo, ma vorrei essere chiaro tenendo conto del contesto internazionale dei mercati finanziari, guarda con attenzione alle iniziative che il settore bancario porrà in essere, o sta ponendo in essere, per attenuare la divergenza tra l'aumento del margine di interesse sui crediti erogati e quello sui rendimenti dei conti correnti, al fine di garantire condizioni più vantaggiose - oserei dire più eque - per le famiglie. ringrazio il signor Ministro. Sono molto soddisfatto di sapere che la questione è all'attenzione che merita da parte del Ministero, perché si tratta di un problema veramente serio per di cittadini italiani e di famiglie. Se posso permettermi, aggiungo un suggerimento. In tema di *moral suasion* con le banche, che è uno degli ambiti che competono al Governo, magari si potrebbe spontaneamente, mi verrebbe da dire - per chi volesse mantenere il tasso variabile, la trasformazione del mutuo a rata fissa, più che a tasso fisso. perché il mutuo a rata fissa consente di evitare le cattive sorprese di un aumento. Sappiamo che, se il cittadino non riesce a pagare, poi non solo non paga l'incremento, ma non paga Quindi, è interesse anche della banca essere saldati per il mutuo, ma si allunga o si accorcia, a seconda del movimento dei tassi, la durata residua del mutuo, evitando così di impattare decisamente sui conti. La ringrazio, signor

lasciasse Londra e naturalmente Milano è stata la candidata ideale per quella posizione, essendo l'Italia una delle più grandi potenze dal punto di vista farmaceutico. Stiamo quindi aspettando finalmente che questa terza sede, che era prevista a Londra, possa arrivare a Milano. In realtà, la trattativa è stata lunga, ma recentemente si è cominciato a temere che il Governo italiano potesse accettare di ottenere una sede a Milano, ma svuotata dalle sue principali competenze. In particolare, il timore era che si perdessero quei brevetti sui cosiddetti *supplementary protection certificate*, i

Quindi, a questo punto, ho una serie di domande da farle. Prima di tutto: a che punto siamo? Verrà la sede a Milano, come lei ha annunciato? È deciso definitivamente, oppure no? La seconda cosa, assolutamente fondamentale, è capire quali competenze verranno a Milano. L'American chamber of commerce in Italy, che si è molto spesa per la sede del TUEB a Milano, anche perché le industrie farmaceutiche americane sono molto interessate al mercato italiano, ha affermato che, se dovesse succedere che le competenze fossero tagliate, si tratterebbe non di un bicchiere mezzo pieno, ma soltanto di alcune gocce d'acqua. L'enorme potenzialità e l'enorme opportunità per Milano di avere questa sede sarebbero dunque sostanzialmente svuotate. Ovviamente, quindi, vorrei sapere quali saranno le competenze. Vorrei sapere anche come sia possibile che ci siamo fatti

stabiliranno degli uffici e assumeranno delle persone e, quindi, cominceranno dal 1o giugno, cioè tra pochi giorni. Quindi, la domanda è anche quando Milano avrà questa sede. Insomma, le domande sono tante. Vorrei che lei ci chiarisse la situazione e, quindi, se il tribunale arriverà a Milano, con quali competenze e da quando.

2023 entrerà in vigore l'accordo sul Tribunale unificato dei brevetti. Si tratta di una tappa importante per la creazione di un sistema brevettuale europeo, che tuteli e promuova l'innovazione e la competitività italiana sui mercati esteri. Il Governo ha portato avanti un'azione diplomatica per sostenere la candidatura di Milano a ospitare una delle sedi della divisione centrale del Tribunale, che prima della Brexit era destinata a Londra. Grazie a questo intenso lavoro, l'Italia ha raggiunto, la scorsa settimana, un'intesa con Francia e Germania, che prevede l'assegnazione a Milano di una sezione della divisione centrale del Tribunale. impegno che il ministro Colonna mi ha appena ribadito nel corso del nostro colloquio, che si è concluso un'ora e mezza fa. L'accordo dovrà ora essere formalizzato dal comitato amministrativo del Tribunale, che si riunirà entro la fine di giugno. La partita negoziale è stata complessa e l'esito tutt'altro che scontato. Il Governo l'ha affrontata in una logica di sistema e con pragmatismo negoziale. Con questa intesa, il Governo ha raggiunto gli obiettivi che si era prefissato: in primo luogo, una rapida decisione per istituire la sede di Milano e renderla operativa in tempi certi; luogo, competenze adeguate in settori importanti per il tessuto industriale del nostro Paese; in terzo luogo, garanzie per il corretto funzionamento della sede di Milano. Abbiamo così evitato che il Tribunale cominciasse a funzionare a regime su due sole località, senza una decisione sulla terza sede, una soluzione transitoria che sarebbe potuta diventare, molto probabilmente, permanente. Le competenze assegnate alla sede di Milano riguardano comparti particolarmente rilevanti per i nostri interessi nazionali, come il settore farmaceutico, la moda e la filiera agroalimentare. Chiederemo inoltre un attento monitoraggio sul funzionamento della sezione di Milano. In caso di sbilanciamento rispetto all'attività delle altre sedi, il Governo si attiverà per ottenere un riequilibrio anche prima dei sette anni previsti per la revisione dell'accordo. Si tratta di un risultato significativo non solo per Milano, ma anche per tutto il Paese, con ricadute positive sull'economia; un nuovo impulso alla competitività e alla capacità di innovazione delle imprese italiane, con contributo al rafforzamento delle nostre esportazioni, uno degli obiettivi prioritari del mio mandato. È un segnale importante che ieri in Commissione politiche dell'Unione europea, proprio qui al Senato, tutti i Gruppi politici si siano espressi a favore di questa scelta del Governo, sottoscrivendo e approvando all'unanimità una risoluzione. Il sostegno trasversale del Parlamento rafforza l'azione dell'Italia in Europa ed è con il gioco di squadra che si ottengono i risultati. È molto importante che il Governo abbia il sostegno del Parlamento, perché il Governo da solo, signor Ministro, non ce l'ha fatta. Io sono molto insoddisfatto di questa sua risposta, perché lei non mi ha detto da quando parte il Tribunale di Milano e non mi ha detto quali sono le sue competenze. In particolare,

perché potrà succedere che sullo stesso prodotto ci siano molti brevetti, uno con l'SPC, uno con la chimica e uno con la farmaceutica; ci si troverà a dover andare in tre diverse sedi del Tribunale. E questo porterà le imprese quasi a ripudiare il sistema che è stato creato, che era invece molto utile. invece molto utile. Inoltre, il comitato amministrativo non ha la competenza di ripartire le competenze, signor Ministro, perché può soltanto stabilire che tutte le competenze di Londra vadano a Milano. Non può cambiare il trattato - per capirci - e tra l'altro proprio il fatto che a Milano arrivi soltanto una parte delle competenze a chiederle: perché quelle competenze potevano stare tutte insieme a Londra e adesso che arrivano a Milano devono essere spacchettate e devono andare a Francia e Germania? Caro ministro Tajani, ho la grande preoccupazione che questo sia l'ennesimo sintomo - lo pagherà la città di Milano e pagherà l'Italia - del nostro isolamento in Europa, perché casualmente chi sono i Paesi che prendono le competenze di Milano? Sono Francia e Germania. Se il suo Ministero non ratifica il MES, se il suo Ministero non ratifica il CETA, lei si immagina di trovare una collaborazione da parte dei nostri alleati europei? Questo è il risultato del vostro isolamento e della vostra politica estera, che soprattutto in sede europea lascia molto a desiderare per l'interesse del Paese.

Signor vice presidente del Consiglio e ministro degli affari esteri Tajani, l'alluvione che ha colpito nelle settimane dal 2 al 17 maggio varie zone dell'Emilia Romagna ha provocato vittime tra la popolazione e grandi danni al territorio il cuore agricolo e industriale della Romagna, con migliaia e migliaia di piccole e medie imprese che hanno subito danni ingenti, ancora in via di quantificazione, e anche una paralisi delle attività. La Regione, le associazioni d'impresa e delle professioni, gli istituti bancari, il terzo settore, i sindacati tutti hanno sottoscritto una dichiarazione congiunta che dettaglia le esigenze del territorio per far fronte alle emergenze e per gettare le premesse per una ripartenza delle attività produttive. Nella dichiarazione c'è anche la richiesta di approntare immediatamente un piano di ristori e di risorse da destinare, oltre che alle famiglie, alle imprese colpite da questi eventi. Tra le richieste vi è quella di contributi a favore delle attività produttive aventi sede e unità produttive nei Comuni interessati dagli eventi calamitosi e che abbiano subito un grave pregiudizio

esportazioni e al successo del *made in Italy* nel mondo. Gli interroganti quindi chiedono al Governo, in particolare al ministro e vice presidente del Consiglio Tajani, quali misure si intendano adottare da parte del Governo per sostenere le attività delle imprese esportatrici delle aree colpite dall'alluvione e per assicurare la loro rapida ripartenza, fondamentale non solo per quel territorio, ma per tutta l'economia italiana. PRESIDENTE. Il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, onorevole Tajani, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, Il Governo si è immediatamente attivato per dare risposte concrete alle popolazioni colpite dalle alluvioni: è stato approvato un decreto da 2 miliardi di euro per i primi interventi. Quattro ore dopo la conclusione del Consiglio dei ministri, ero a Forlì per illustrare alle amministrazioni locali, alle imprese, ai sindacati e ai cittadini come si potevano utilizzare i fondi messi a disposizione dal Governo, in modo particolare quelli legati al coordinamento del mio Ministero. Proprio per dare risposte concrete, ho chiesto ai vertici dell'Agenzia ICE e di Simest, Sace e Cassa depositi e prestiti di essere Nell'area colpita dal disastro, nelle province di Forlì, Cesena e Ravenna, quasi 25.000 imprese occupano 270.000 persone e fatturano 70 miliardi; moltissime hanno una forte proiezione internazionale. Le aziende esportatrici potranno contare su un pacchetto di misure di 705 milioni di euro predisposte dal Ministero degli affari esteri con Simest e Agenzia ICE. Nell'immediato, 300 milioni di euro di ristori a fondo perduto compenseranno le perdite materiali subite e le riduzioni di reddito causate dalla sospensione delle attività. Non vogliamo certo limitarci all'emergenza. Per la ripartenza abbiamo riservato 400 milioni di euro del Fondo 394 gestito da Simest per finanziamenti con tassi agevolati e a fondo perduto del 10 serviranno a ripristinare i beni danneggiati e a finanziare progetti di internazionalizzazione. Alla misura potranno accedere, senza presentare garanzie, le imprese esportatrici delle aree alluvionate, ma anche quelle che, pur non esportando direttamente, operano nella stessa filiera. In aggiunta, i rimborsi dei finanziamenti già attivi sul Fondo 394 vengono sospesi per dodici mesi. Sul Fondo ICE, nell'ambito di un pacchetto di oltre 5 milioni di euro, l'Agenzia offrirà gratuitamente i servizi della propria rete nel mondo, un modulo espositivo nelle fiere all'estero, attività promozionali anche di *e-commerce*, pubblicità, consulenza e formazione all'*export*. Sace ha varato una serie di iniziative in ambito credito, liquidità e cauzioni. Penso anzitutto alla moratoria fino a un anno sui finanziamenti garantiti e alla sospensione del pagamento dei premi delle polizze fino al 31 dicembre. A favore di micro e piccole imprese proiettate all'internazionalizzazione, Invitalia propone inoltre un bonus *export* digitale a fondo perduto; il possibile utilizzo va dal riacquisto dal riacquisto di strumenti informatici danneggiati all'assistenza per *marketing* e vendita attraverso l'*online*. Sono strumenti concreti che le imprese potranno attivare con facilità. Esse avranno inoltre a disposizione un indirizzo di posta elettronica per chiarimenti su come accedere alle misure previste. È già aperto da due giorni e lo ripeto perché possiate diffonderlo:

Siamo vicini alle famiglie che hanno perso i propri cari e daremo tutto l'aiuto possibile a chi ha visto distrutto il lavoro di una vita. Come Ministro degli affari esteri e del commercio internazionale sento la responsabilità particolare di restituire, alla seconda Regione esportatrice d'Italia, il dinamismo che la rende famosa e apprezzata nel mondo. L'Emilia Romagna ripartirà subito, più forte di prima, con il sostegno di noi tutti e la tempra della sua gente straordinaria.

rispondeva di un'intesa raggiunta un'ora e mezzo fa: riferire più in tempo reale di così al Parlamento non si può. Quindi, la ringrazio, non solo per la risposta al quesito postole, ma anche per tutta la sua attività politico istituzionale, preziosa per la Repubblica italiana.